*dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro della cultura e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:* "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"

come noto, il 17 luglio scorso la Commissione europea ha inviato al Governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

in tema di previdenza, assistenza e maternità e anche in ordine a un decoroso trattamento economico che sia corrispondente all'alta funzione che essi svolgono. Pertanto, signora Presidente, le chiedo ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, lei inviti il ministro Cartabia a riferire con urgenza al Parlamento e a quest'Assemblea

La relatrice, senatrice Modena, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 11-*octies*, reca misure di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento di costi fissi. Si segnalano, in particolare, alcune disposizioni. L'articolo 1, commi 1 e 4, riconosce e disciplina un contributo a fondo perduto, "ulteriore" rispetto a quelli previsti dai provvedimenti precedenti, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (26 maggio 2021). I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi dal 16 al 27 disciplinano un diverso contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti indicati nei commi 16 e 17. Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19». L'articolo 1-*bis* abroga il comma 9 dell'articolo 6-*bis* del decreto legge n. 137 del 2020 (decreto-legge ristori), pur mantenendo ferma la detassazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi ivi elencati, in quanto ricompresi nel disposto dell'articolo 10-*bis* del medesimo decreto-legge ristori. l'erogazione dei contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il massimo di spesa alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore cosiddetto Horeca. L'articolo 1-*quater* incrementa di 60 milioni di euro per 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore. L'articolo 1-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza negli anni 2020 e 2021, sempre in ragione dell'emergenza Covid. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali, l'adozione di dispositivi di protezione personale per ospiti e operatori e l'adeguamento strutturale dei locali. L'articolo rimodula i tempi di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente di riscossione. 1-*septies* contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione, istituisce al primo comma nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati sono stati aggiunti tre commi ulteriori che incrementano di 50 milioni per il 2021 il fondo destinato alle perdite derivanti dall'annullamento, seguito all'emergenza da Covid-19. L'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge sostegni per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, L'articolo 3-*ter* autorizza la spesa di 35 milioni per il 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano e Cortina 2026. L'articolo 4 proroga al 31 luglio lo specifico credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, previsto per le imprese turistiche ricettive, le aziende di viaggio e i *tour operator* che hanno una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. L'articolo 4-*ter* esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione si applica nel caso in cui, per il 2021, la convalida sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede di corrispondere un ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall'agevolazione. L'articolo 5-*bis* conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo complessivo di 1.200 milioni di euro anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe nel settore elettrico, fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e per il terzo trimestre dell'anno 2021. L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, oppure dalle restrizioni. L'articolo 7 reca una serie di misure rivolte al sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte, tra le quali il rifinanziamento di 160 milioni di euro del fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide, gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane o suburbane. Include inoltre i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator*, tra quelli il cui pagamento è coperto dalla *tax credit* vacanze. L'articolo 7-*bis* consente l'utilizzabilità del credito riconosciuto per il pagamento dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale anche per il pagamento dei pacchetti turistici. L'articolo 8 modifica la condizione del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Rifinanzia inoltre di 120 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo istituito nello Stato di previsione del MEF da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, in particolare le imprese esercenti le attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme, derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito di imposta e il debito iscritto a ruolo. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. I commi successivi modificano la disciplina delle attività che sono svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il comma 1-*septies* stabilisce che i fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, verificatisi nell'agosto del 2017 a Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati. Il comma 3 di questa disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta *plastic tax*, ovvero dell'imposta di consumo dei manufatti con singolo impiego. Abbiamo poi anche un termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili verso i soggetti che non abbiano provveduto a fare delle dichiarazioni al catasto edilizio urbano per i terreni che sono ubicati nel settore del sisma la Camera ha anche ampliato la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi. Il 9 comma-*bis* proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti che attengono la Tari da corrispondere nel 2021.

Presidente, ringrazio lei che mi lascia sedere tra i banchi della minoranza, dove c'è meno dispersione e meno difficoltà a parlare, visto che lì c'è un continuo viavai e per me è quasi impossibile intervenire. Quindi, resto comodamente nel nostro nido d'aquila

il pensiero, il convincimento, le motivazioni e qualsiasi contributo che l'opposizione può darvi. Lo dimostrano i fatti. Ricordo da spettatore, da sindaco,

lagnava giustamente per il ricorso ossessivo e compulsivo al voto di fiducia. Quella stessa minoranza oggi è maggioranza e non si vergogna nemmeno più

e poi il provvedimento arriva blindato nell'altra Camera, dove il relatore di minoranza ha un ruolo assolutamente pleonastico; fa un esercizio di retorica inutile dal punto di vista dell'incidenza sul provvedimento, ma utile a ricordare una cosa a tutti qua dentro. Vedo le teste che si abbassano perché tanti hanno fatto parte dell'opposizione anche in questa legislatura e dicevano le stesse cose che dico io. Oggi, invece, sono costretti a farsi andar bene anche questa prassi ormai consolidata che svilisce o vorrebbe svilire il ruolo delle opposizioni e renderle Invece crediamo che anche solo il fatto che esistiamo sia per voi una fonte di grandissimo imbarazzo, perché siamo qui a ricordarvi che la democrazia è un'altra cosa, siamo in pochi

che voi avete introdotto per giustificare i vostri ritardi atavici nell'emanare i provvedimenti che poi devono "correre" in Aula, pena la loro decadenza. Credo che la vergogna che dovreste provare basterebbe oggi al relatore di minoranza per dire che si sta discutendo di un provvedimento di 40 miliardi con dei tempi

tutto quello che viene discusso in questa sede e che viene proposto da persone democraticamente elette è importante, ma forse non è una priorità rispetto invece a quello che ci chiedono le imprese, tanti operatori, le partite IVA, che vorrebbero

perché così riuscirete a fare un po' di campagna elettorale e proseliti tra quelli che pensate costituiscano ormai il vostro elettorato di riferimento, che in realtà sempre più si stanno rendendo conto di quanto bisogna uscire dai temi ideologici e simbolici per entrare nei temi pratici, concreti e che afferiscono ai diritti della persona in senso generale, non solamente di una parte di diritti di una parte delle persone. I diritti sono inalienabili, ma appartengono a tutti; non esistono persone che hanno più diritti degli altri, non esistono nemmeno persone ghettizzate più delle altre. La persona è una e di queste persone dovremmo occuparci come con questo decreto. la Camera ha approvato mercoledì scorso, 14 luglio, che oggi arriva al Senato blindato, come ho già avuto modo di spiegare, è un decreto che è sostanzialmente la continuità dei Governi che hanno preceduto il Governo Draghi. La metodologia è la stessa: il contributo a pioggia, la scarsità di visione, la mancanza di una strategia d'uscita da questa pandemia. Già il fatto che dopo un anno e mezzo si stia ancora parlando di emergenza dimostra il fallimento di un anno e mezzo di politiche dell'emergenza, perché un'emergenza ha un tempo limitato e contingentato, la visione e il futuro dovrebbero avere un tempo decisamente diverso. In realtà, già dicendo che è un decreto d'emergenza implicitamente abdicate al vostro ruolo e manifestate la vostra palese incapacità di risolvere i problemi di questa Nazione. Ve lo diciamo da opposizione patriottica. Qui non siamo mai venuti senza una proposta, abbiamo sempre aggiunto alla protesta la proposta ed è per questo che fuori, nel mondo reale, questo stando ai sondaggi è il primo partito della Nazione, mentre qui dentro è ridotto ad uno spicchio senza la possibilità di incidere sui provvedimenti. Non è perché noi, come ha fatto una parte dell'emiciclo nella scorsa legislatura, abbiamo raccolto i mal di pancia di tutti, perché in questa legislatura abbiamo detto chiaramente qual era il nostro pensiero e intorno a questo pensiero concreto

che hanno avuto un po' più di tempo, hanno fatto un grandissimo lavoro; penso al capogruppo Trancassini, ma chiunque si sia alternato in Commissione bilancio ha tentato di migliorare questo provvedimento.

Se si vota nelle maggiori città italiane non c'è alcun motivo per cui non si possa votare anche per questo Parlamento. Vi accorgerete che probabilmente quel consenso che qua dentro, in maniera bulgara, credete di esercitare, al di fuori, tra la gente non esiste. *(Applausi)*.

chiara ed esaustiva relazione di minoranza del collega De Carlo, vorrei dire innanzi tutto che la sottoscrivo. La sottoscrivo non tanto e non solo come collega e amico del sindaco e senatore De Carlo, ma come cittadino che, di fronte a tante oggettive verità, non può che essere condiscendente. Presidente, credo di aver affrontato con una certa durezza,

Presidente, così come alla presidente Casellati e a tutti i Presidenti di Commissione, l'appello che ho espresso al presidente d'Alfonso e al presidente Pesco nelle Commissioni competenti alle quali ieri ho partecipato. Mi rivolgo agli organi che rappresentano le istituzioni democratiche della Repubblica, i quali hanno il dovere - lo sottolineo - di tutelare la Costituzione. Siamo di fronte a un'inaccettabile violazione della Costituzione italiana. Siamo di fronte a un monocameralismo di fatto, dimenticando peraltro che c'è un *referendum* che, rappresentando gli italiani, ha bocciato la riforma della scorsa legislatura. Quindi, a prescindere dalle convinzioni di ciascuno, siamo tenuti, in quanto rappresentanti del popolo, a rispettare la Costituzione. Eppure, ciò non accade perché ormai il Parlamento sta viaggiando su due binari: quello della decretazione d'urgenza ma sappiamo benissimo che, se è urgenza, non può essere ordinaria, almeno per terminologia e vocabolario - e quello del voto di fiducia. Dal momento che questa è una ripetuta e ormai consolidata violazione della Costituzione, chiedo che le cariche istituzionali che rappresentano il Parlamento tutto si rivolgano - e lo chiedo formalmente - al Presidente della Repubblica. È inaccettabile che si proceda violando la Costituzione. È inaccettabile che provvedimenti che investono miliardi vengano di fatto approvati da una sola Camera, che vedano in questo caso il Senato completamente delegittimato e costretto a un mero voto, senza poter toccare palla, come si suol dire, senza poter modificare alcunché. È inaccettabile secondo buonsenso, ma soprattutto illegittimo perché contro la Costituzione italiana.

a indicare un decreto attuativo realizzato sui 41 previsti dal decreto sostegni-*bis*; su 149 sono i decreti attuativi realizzati su tutta la normativa Draghi. Che cosa vuol dire cosa vuol dire per chi ci ascolta? Vuol dire che è un po' come andare a spendere dei soldi, ma, anziché tramutarli in atti concreti - perché il decreto attuativo serve a tramutare la norma in qualcosa di concreto - vengono messi e isolati in frigorifero. È un po' come una persona che vuole andare in macchina da Trento, la mia città, a Roma e fa il pieno di benzina o di gasolio; però, invece di mettere il carburante nel serbatoio, lo mette nelle taniche e lo tiene nel baule della macchina, che dunque non arriverà mai a Roma. Quindi, i miliardi che stiamo investendo e con i quali ci siamo indebitando sono in gran parte nel frigorifero, nel baule della macchina, non finiscono nell'economia, non finiscono nelle tasche delle imprese, degli artigiani e dei commercianti.

allora ci sono colleghi - mi rivolgo ai colleghi del centrodestra che, insieme a noi, lottavano contro i decreti attuativi - che perseverano perseverano ancora, da una parte, nella decretazione d'urgenza e, dall'altra, nel prevedere nelle norme decreti attuativi *ad abundantiam* che poi non si trasformano, come dai numeri che ho letto, in atti concreti?

Entro poi nel merito perché certamente, come ha detto il collega De Carlo, noi siamo una forza fieramente di opposizione, ma altrettanto orgogliosamente e fieramente di proposta.

perché, a distanza di un anno e mezzo dall'inizio della pandemia (diciotto mesi), continuiamo a lavorare sull'emergenza? Perché da diciotto mesi siamo ancora qui a parlare di sostegni e di ristori e di fatto non solo non li traduciamo in atti concreti, come ho detto prima, ma non abbiamo ancora la benché minima sostanza di politiche costruttive attive? Blocchiamo i licenziamenti, ma dove sono le politiche del lavoro? Fratelli d'Italia ha proposto un regime premiale per le imprese che non licenziano e che assumono: perché non ci rispondete? Perché il Governo non cerca di passare dal blocco dei licenziamenti ai regimi premiali per chi accresce l'occupazione, per quegli imprenditori che tengono duro, mantengono i dipendenti e magari ne assumono di nuovi? Ecco le proposte concrete per andare oltre l'emergenza, per costruire un percorso e un futuro. Per quanto fisco, sono poco più di 20 miliardi i soldi che - tra il decreto sostegni e il decreto sostegni-*bis* - vanno alle imprese. Il centro studi della CGIA di Mestre lo ha dimostrato oggettivamente:

le imprese, gli artigiani, i cittadini, cioè quelle persone che avete tenuto chiuse, nonostante tanta contrarietà, anche da parte nostra, e che hanno dovuto però continuare a pagare i contributi, le imposte, gli affitti, i costi fissi.

che da settimane, da mesi, giaceva la legge sull'equo compenso; adesso sembrava ad un passo, ma a tutt'oggi alla Camera non risulta in votazione. Abbiamo il disegno di legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti. Mi rivolgo anche alla vice ministro Castelli, qui presente, e chiedo che si decida di dare una mano a quei professionisti che non vogliono assistenzialismo, ma vogliono essere sostenuti quando purtroppo capitano loro infortuni e malattie. Presidente, è che si rispetti la Costituzione, che il Presidente della Repubblica ponga fine alla delegittimazione delle Istituzioni e delle regole democratiche e che tutte le forze politiche presenti in Parlamento passino dall'assistenzialismo e dall'emergenza alle fasi costruttive ed operative nell'interesse del Paese.

impegnarci a valutare l'opportunità di vaccinarci. *(Applausi)*. Lo dico perché esco da un isolamento volontario. Lasciando ampia libertà, valutiamo però l'opportunità.

Ci sono però alcune criticità che dobbiamo evidenziare. La prima: non dobbiamo abituare il Paese, l'economia e il sistema produttivo alla politica dei sostegni, alla politica degli aiuti.

Ho la sensazione che il Paese si stia abituando troppo ai sussidi economici che arrivano e che non potranno continuare Lo ha richiamato anche il governatore della Banca d'Italia Visco in occasione delle conclusioni finali. È stato chiaro: non si può andare avanti vivendo di sussidi. Io so che c'è l'attenzione del Governo, del suo Presidente, delle forze della maggioranza e ci sarà anche lo stimolo dell'opposizione per far sì che si possa uscire in fretta da questa situazione. che avremo superato l'emergenza sanitaria e saremo usciti dall'emergenza economica, normale conseguenza della prima. Mi auguro e ci auguriamo che questo sia l'ultimo intervento che facciamo in termini di sostegni perché ciò vorrà dire che la crisi in parte è stata superata. Ci sono moltissimi aspetti del decreto-legge sostegni*-bis* che ci piacciono. Ricordo, tra tutti, anche l'accordo e la mediazione intelligente che è stata trovata sugli ammortizzatori sociali, sullo sblocco dei licenziamenti per quei settori economici, fortuna che ci sono, che stanno andando bene, il manifatturiero e l'edilizia. manifatturiero e l'edilizia. Non ce ne vogliano i colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma ci piacerebbe, per esempio, che i fondi cospicui destinati al reddito di cittadinanza fossero convertiti a fondi per ridurre le tasse sul lavoro, per creare opportunità di lavoro, anziché favorire politiche sociali secondo noi poco positive. *(Applausi)*. Sblocchiamo le tasse sul lavoro se vogliamo ripartire; sblocchiamo le tasse sul lavoro se vogliamo passare da una politica sostenuta e sussidiata ad una politica che vive e si sostiene con le proprie gambe. Attenzione, è un decreto-legge che ha una valenza in termini economici e finanziari di una legge di bilancio pre-Covid.

sono tutte manovre a debito e i debiti, prima o poi, bisogna riportarli a casa e ripagarli. O il Paese cresce, e allora ha la capacità e la forza di poter ripagare il debito, o attualmente

servono debiti buoni e riforme buone. Questo è compito della maggioranza, del Parlamento: approvare in fretta le riforme per portare a terra il prima possibile i fondi del PNRR. Signora Presidente, lo dico sempre e lo ripeto anche questa volta: un sistema del genere porta la nostra economia a far sì che chi sta bene stia meglio e chi sta male stia peggio. Attenzione, perché dal punto di vista della tensione sociale questa è una bomba che abbiamo sotto di noi.

per esaminarlo anche qui in Senato. Ovviamente siamo in un momento di emergenza, ci sono delle regole ben precise dettate dai regolamenti e dalla situazione politica, per cui spesso

grazie a tutto e che sarebbe importante ascoltare anche per riuscire a comprendere come loro hanno lavorato. Riporto stralci del suo intervento: «un lavoro, devo dire, svolto in sinergia, un lavoro di Commissione che ha portato a integrare e modificare le misure, estendendone il campo a molte realtà in crisi che erano state escluse dai contributi e aiuti concreti. Questo è stato il tema che ha affrontato la Commissione, con emendamenti comuni, emendamenti condivisi da tutti i movimenti e partiti politici». Questo è un dato importante, lo dice Massimo Bitonci, lo dice il relatore del provvedimento, che ci dà contezza di come sono andate le cose. Un decreto che immette 44 miliardi complessivi nel mondo reale: aiuti alle imprese, al lavoro, ai giovani, alla salute, al territorio. Due volte una legge di bilancio che, se sommato al "Sostegni", supera i 70 miliardi di misure atte ad aiutare il sistema produttivo, le famiglie, le associazioni, il volontariato, per superare la grave crisi economica che ha colpito la nostra Nazione durante la pandemia. Alla fine del 2019 l'economia italiana presentava già evidenti segnali di stagnazione; poi, a partire da fine febbraio, il dilagare dell'epidemia Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo precedente hanno determinato un impatto profondo sull'economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento, consumo e funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali.

14 miliardi di erogazioni dirette con un'importante novità: si introduce un correttivo che tiene conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite e dei costi fissi di esercizio per le aziende con volume d'affari aumentato da noi (cioè dalla Lega) di oltre 15 milioni. Dalla Lega un vero sostegno l'Italia: abbiamo prorogato al 15 settembre il saldo e acconto delle tasse di giugno e luglio, una boccata di ossigeno e di liquidità per le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti. Oltre a questo, abbiamo ottenuto un'ulteriore proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente di riscossione: 163 milioni di cartelle giacenti per 18 milioni di italiani e un ulteriore differimento della rateizzazione del pagamento della rottamazione-*ter* e saldo e stralcio entro l'anno in corso». Non basta, però, come sostiene Bitonci «pensare a misure strutturali, deflattive del contenzioso, una nuova pace fiscale che cancelli definitivamente quanto non è più esigibile, non parlo dei furbetti di turno che vanno stanati, ma di aziende» e la Lega continuerà a ripeterlo. pensato ai dimenticati dai "ristori", al turismo, che produce il 13 per cento del PIL nazionale, agli hotel, ai ristoranti, ai bar, al settore del *wedding*, agli eventi, con 70 milioni, alle fiere nazionali, che sono ancora oggi luoghi messi a disposizione per la vaccinazione al terzo settore, case di riposo, aree termali, centri riabilitativi, alle guide turistiche e agenzie di viaggio, al settore delle crociere, bus turistici, città d'arte, impianti di risalita sciistici minori, all'editoria, al ristoro per attività «Non ci siamo dimenticati dei connazionali terremotati e delle aree colpite da sisma, estendendo al 31 dicembre il credito d'imposta per le imprese che effettuano gli investimenti e per chi ha il coraggio e la forza di fare ancora impresa in quelle zone gravemente colpite, come per i contributi per i nostri agricoltori, colpiti pesantemente, oltre che dalla pandemia, anche da gelate, alluvioni e calamità naturali. Per lo sport abbiamo destinato 112 milioni di euro a fondo perduto per gli operatori del settore, per la gestione e manutenzione delle piscine e per gli interventi infrastrutturali su impianti sportivi per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026». Non si sono dimenticati neanche della sanità e del sociale, delle cure palliative, del Fondo per gli istituti oncologici e pediatrici e dell'inclusione e del finanziamento delle scuole d'infanzia paritarie. PRESIDENTE. La prego di

nel corso del 2020 sono state introdotte, per fronteggiare l'emergenza economica causata dalla pandemia da Covid-19, forme di sostegno che hanno superato, in termini economici, i 100 miliardi una cifra corrispondente all'incirca al 7 per cento del PIL nazionale. Quest'ultimo decreto-legge, che ci apprestiamo a convertire in legge, mette sul piatto ulteriori 45 miliardi di euro, distribuiti capillarmente a tutte le categorie economiche che hanno subito pesanti ripercussioni nell'emergenza epidemiologica. Questo provvedimento corrisponde a una vera e propria legge di bilancio, un imponente pacchetto di misure necessarie e doverose per rimaneggiare gli eventi negativi e disastrosi della pandemia. Considerate le moltissime modifiche e novità che sono state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, desidero soffermarmi soltanto su alcuni suoi aspetti. Il decreto-legge introduce un importantissimo pacchetto di misure economiche a sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali ad esso legate, che in quest'ultimo anno hanno subito fortemente, sono state danneggiate e necessitano assolutamente di rimettersi in moto. infatti è un Paese che vive di turismo, noto in tutto il mondo per le sue immense bellezze naturali e culturali. Il nostro Paese è, senza alcun dubbio, una delle mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le sue condizioni climatiche, climatiche, naturalistiche, socioculturali, archeologiche, termali ed enogastronomiche. Dobbiamo però consentire agli operatori del settore di avere delle solide basi su cui sostenersi e poter affrontare al meglio questa complessa stagione turistica. un pacchetto importantissimo, che introduce ad esempio 150 milioni di euro, per l'anno 2021, per il fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici e, ancora, un'indennità di 1.600 euro a favore delle diverse categorie di lavoratori del settore e altri interventi a sostegno delle strutture alberghiere e ricettive. Tra queste misure di rilevante interesse c'è sicuramente quella legata ai bus turistici, per i quali è stato introdotto uno stanziamento di quasi 10 milioni di euro, da destinare come contributo a fondo perduto per l'intero comparto. Un altro punto sul quale vorrei soffermare l'attenzione della discussione riguarda le misure pensate per il commercio sulle aree pubbliche, il cosiddetto commercio ambulante, uno dei principali pilastri della distribuzione italiana, in grado di dare lavoro ad oltre 190.000 imprese e a più di 217.000 addetti, con un fatturato complessivo di 11,1 miliardi di euro. Anche questo comparto sta vivendo una crisi gravissima e già 6.000 piccole aziende e attività ambulanti hanno cessato la loro attività dal giugno 2019 al giugno 2020. Con l'articolo 56-*bis* si attribuisce ai Comuni la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, entro il termine dei novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. La disposizione determina di fatto la possibilità di prorogare il procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e si pone l'obiettivo di ridare certezza ad un settore, che negli ultimi anni abbiamo già visto

altro importante traguardo riguarda il rifinanziamento di 120 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo a sostegno di alcune attività particolarmente colpite dall'emergenza, ovvero quelle degli eventi e dei *catering*, dei parchi tematici e degli acquari, dei parchi geologici e dei giardini zoologici, del *wedding* e delle attività commerciali come la ristorazione, che operano all'interno dei piccoli centri dell'entroterra. L'articolo 1-*ter* pone attenzione alla filiera dell'Horeca, ovvero alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste, di cerimonie, del settore dell'*hotellerie*, del *restaurant* e del *catering*, con l'erogazione di contributi a fondo perduto, per un importo complessivo di 60 milioni di euro. Tale filiera rappresenta oltre 60.000 lavoratori e 3.800 aziende, la maggior parte a conduzione familiare, sparse sull'intero territorio nazionale, con micro-imprese familiari patrimonialmente deboli e inconsistenti Le misure di ristoro alle imprese non sono riuscite a contenere gli ingenti danni subiti dal comparto della distribuzione, che ha visto calare il fatturato di ben 7 miliardi di euro, dai 17 miliardi del 2019 ai 10 miliardi di euro del 2020, con un crollo del 37,6 Dobbiamo essere consapevoli del fatto che, nonostante le misure adottate, sono necessari ulteriori sforzi per risollevare le aziende e gli operatori del settore, che hanno esplicitamente chiesto aiuto al Parlamento, per contrastare la crisi economica che da oltre un anno li li sta colpendo duramente. La distribuzione *food and beverage* non è stata chiusa. Di fatto, con i precedenti decreti sussidi, gli operatori sono stati esclusi per la questione del codice Ateco, che li ha mantenuti aperti, ma ma il loro settore non aveva possibilità di operare, perché la ristorazione e tutti i settori dell'accoglienza erano praticamente chiusi.

dal rinvio delle fiere e dei congressi su tutta l'area nazionale. Si tratta di un problema che ha colpito in maniera forte anche la logistica, il trasporto e l'allestimento, che hanno operato all'interno di questo settore. Spero che questo sia l'ultimo decreto-legge necessario per fornire sostegni e sussidi alle tante categorie economiche colpite duramente dall'emergenza epidemiologica. I segnali di ripresa sono dovuti soprattutto all'ottimo andamento della campagna vaccinale, ma è su questo che il Paese non deve demordere e deve ancora migliorare. La migliore misura per il rilancio dell'economia e per il ritorno alla completa normalità al momento è solamente la strada della vaccinazione, che sarà l'unica soluzione che ci porterà fuori dalla situazione che stiamo vivendo in questo momento. *(Applausi)*. Queste misure, unitamente alla campagna vaccinale, ci hanno concesso di portare tutto il Paese e tutta la nostra penisola in zona bianca (con conseguente apertura di bar, ristoranti e musei) e di riacquistare dei piccoli spazi di libertà che sembravano normali fino ad alcuni anni fa, ma che adesso sono molto difficili da raggiungere. È importante continuare su questo percorso, ma anche rimanere assolutamente prudenti e fare molta attenzione, perché in questa situazione è sottilmente labile l'area su cui ci stiamo muovendo; tutta la popolazione deve essere estremamente attenta in questo momento. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà. rappresentante del Governo, colleghi, ieri in 6a Commissione (Finanze) si è sviluppato un interessante dibattito trasversale tra i commissari senatori a riguardo del sistema procedurale di questi mesi direi anche di questi anni). Si sta verificando uno scollamento tra Parlamento e Governo nel modo di procedere all'approvazione dei decreti-legge,

Praticamente, gli emendamenti che vengono presentati nella seconda Camera, che troppo sovente è il Senato (al di là della consuetudine dell'incardinamento a rotazione tra le due Camere), pongono questi problemi: ci sono degli emendamenti di ordine normativo, che quindi possono essere esaminati e possono essere positivi per la soluzione dei problemi, e ci sono emendamenti di spesa che patiscono la situazione di difficoltà, che il MEF esprime con un parere negativo. Ci sono delle aggravanti in questa situazione, perché - lo dico in tono costruttivo, sia chiaro, seppure in maniera ferma ci sono settori che non sono ancora partiti e che incontrano delle difficoltà e ce ne sono altri che faticano a partire. Ci solo delle situazioni in cui i sostegni, di cui al decreto-legge che approveremo oggi o domani, non hanno avuto riconoscimenti per una serie di motivi, giusti o sbagliati (dimenticanze, valutazioni). Ci sono dei settori che hanno patito maggiormente la situazione. Faccio un esempio che non è banale: le sale e le orchestre da ballo hanno chiuso per prime e apriranno per ultime, ma sono settori che raggruppano decine di migliaia di persone tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Come ho detto in un mio intervento precedente su uno dei tanti provvedimenti economici, pensavo che, superata la questione dei codici Ateco, si potesse arrivare (è una provocazione, ma non tanto, perché si tratta di prendere una decisione) al punto che i sostegni andassero a tutte le partite IVA, senza domanda, (è successo in tanti Stati) eliminato così burocrazia pubblica e privata. Faccio un esempio preso dagli emendamenti che ho presentato e che non saranno ovviamente discussi, perché sarà posta la fiducia. Ci sono delle attività che hanno aperto nel 2020, per loro fortuna o sfortuna, subito dopo il primo *lockdown*, perché avevano l'apertura in previsione e avevano fatto degli investimenti e dei contratti. Qual è il fatturato di riferimento di queste imprese,

Gli sfratti sono una punizione per i proprietari. È stata introdotta la norma che permette di non versare l'IVA sulle fatture entrate nei fallimenti a partire dal 19 maggio, ma è probabile che sarebbe stato più giusto

siamo di fronte a un provvedimento importante, ricco di contenuti e soprattutto - come quasi mai abbiamo visto - di concretezza, con la volute e richieste. In quest'epoca ciò è il tipico esempio che mette in evidenza la differenza tra il precedente Governo giallo-rosso e quello attuale, che

in merito all'applicazione dell'IVA sulle operazioni di cessione di selvaggina da parte degli allevatori. Oggi, all'articolo 18-*bis* del provvedimento in esame, si legge

nostro Paese, che in Europa è quello con la più alta concentrazione di fauna selvatica, sono circa 3 milioni i capi allevati e messi a disposizione di circa 2.500 aziende faunistiche e agro-faunistico-venatorie e degli allevamenti,

sono 244 gli ambiti territoriali di caccia, 75 i comprensori alpini, 492 le riserve alpine e 20 i distretti venatori. Bene hanno fatto coloro che hanno avviato lo sviluppo della filiera alimentare di carne di selvaggina, nel rispetto della sicurezza alimentare e dell'ambiente, e bene ha fatto la Regione Lombardia a siglare un apposito protocollo di intesa su questo tema. Si tratta di carni pregiate, come dimostra il forte interesse nazionale dei ristoranti stellati. Si tratta di un settore dell'agroalimentare che merita un razionale intervento del legislatore. Dobbiamo agevolare lo sviluppo del consumo di queste carni anche con la modifica di norme esistenti ma abbondantemente superate. superate. Noi diciamo: meglio le carni della nostra fauna selvatica piuttosto che gli insetti che ci propina l'Europa.

è compreso il riconoscimento del fatto che la fauna selvatica allevata è destinata all'alimentazione. Invito pertanto tutti i colleghi, ma soprattutto il Governo, a chiarire definitivamente che l'aliquota da applicare alla selvaggina allevata è del 10 per cento, come chiesto con la mia interrogazione di due anni fa. Oggi su questo tema - mi rivolgo ai colleghi di Fratelli d'Italia, che mi pare d'aver capito siano intenzionati a votare contro - abbiamo un risultato importante; portiamo a casa un risultato concreto e immediato che aiuta le nostre aziende in questo settore, ma soprattutto apriamo una porta

ringrazio per l'attenzione, ma soprattutto ringrazio chiunque vorrà tenere conto delle cose che ho appena detto, perché inizia un percorso nuovo e credo che sia un percorso sano, anche se di chiara contrapposizione ad alcune proposte alimentari che arrivano dall'Europa.

le pressioni maggiori che si sono riversate sulle strutture ospedaliere proprio in concomitanza con il Covid, che ha creato una situazione di

indagini sotto il profilo genetico molto sofisticate, e incrementando quello che potremmo chiamare il tagliafile - sappiamo quanto è lungo il tempo di attesa

dei pazienti che si sono ammalati di Covid in questo periodo e che potranno sottoporsi, per due anni e senza costi a loro carico, ad un controllo costante e continuo. Si rivolge però anche a quei pazienti che durante questo periodo hanno dovuto soffrire, sotto il profilo psicologico, tutto il disagio derivato dal *lockdown*, quindi dalla limitazione dei rapporti interpersonali e dall'ansia che ne può essere scaturita, compresa l'ansia provocata dalla perdita di opportunità professionali. Adesso stiamo tutti leggendo, con grande compartecipazione, non solo sotto il profilo emotivo, ma anche sotto quello della ricerca di soluzioni, notizie di persone che dovranno affrontare il rischio licenziamento.

un po' depotenziato nel tempo: abbiamo bisogno di nuovi antibiotici. Abbiamo bisogno di una ricerca che vada anche in questa direzione, accanto a quella che riguarda gli anticorpi monoclonali.

ha un'importanza vitale per tutta l'economia del nostro Paese, com'è stato detto bene anche prima. Tuttavia, relativamente al tema sul quale mi vorrei soffermare, l'agricoltura, questo provvedimento vale un miliardo di euro di aiuti diretti.

un sostegno vero, non solo a parole, per l'anello più debole della filiera agroalimentare italiana: il contadino, l'agricoltore, il pescatore, figure straordinarie che anche in questo anno e mezzo di pandemia non hanno mai smesso di lavorare, di sostenere e procurare il cibo e di dare dignità al ruolo di coltivatori e custodi della terra, di pescatori e custodi del mare. Questo lo dobbiamo riconoscere a tutti i nostri produttori. alcune delle misure che abbiamo approvato: noi assegniamo con questo provvedimento ad Ismea 80 milioni di euro, al fine di rafforzare uno strumento importantissimo, quello delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca.

Molti nostri imprenditori non riuscivano a finire gli investimenti perché non potevano cumulare una garanzia con un'ipoteca. Invece ora sarà possibile; abbiamo dato la stessa possibilità offerta alle imprese turistiche e alberghiere.

sono misure concrete anche sul settore zootecnico, che sta soffrendo tantissimo. È in discussione il futuro di generazioni che stanno lavorando per le tensioni del mercato nazionale e internazionale sugli alimenti per il bestiame. Abbiamo incrementato il Fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere di ben 5 milioni di euro, da erogare nel corso del 2021, con aiuti diretti agli allevatori di bovini. Un ulteriore sostegno importante arriva dalla compensazione IVA applicabile alle cessioni di animali vivi (bovini e suini). L'abbiamo innalzata al 9,5 per cento: 28 milioni di euro sono destinati a questa misura importante.

È stato istituito - questo è importantissimo - un Fondo per il sostegno bieticolo-saccarifero con una dotazione di 25 milioni di euro per i produttori italiani particolarmente danneggiati dalla pandemia e dalle riduzioni dei volumi di *export*. Il contributo verrà erogato sulla base delle superfici coltivate. Questo è fondamentale perché andiamo ad aiutare il produttore primario. Viene istituito e finalmente istituzionalizzato il sistema di anticipazione al 70 per cento del pagamento dei premi PAC in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o dalle crisi di alcuni settori. Abbiamo aggiunto a questa disposizione anche le perturbazioni di mercato con la modifica del cosiddetto quadro temporaneo. L'anticipazione viene erogata compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta. poi quella che credo sia la misura più importante del provvedimento. Mi riferisco alle indennità per i lavoratori del settore agricolo che abbiano svolto almeno 50 giornate lavorative per il 2020

Per quanto riguarda poi il tema dei birrifici, che sovente viene ripreso nei vari emendamenti e nelle diverse misure, ma poi naturalmente dalla Commissione bilancio e dal Governo arrivano dei dinieghi, oltre all'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, così come fatto anche per le aziende produttrici di vini, abbiamo riconosciuto finalmente un contributo a fondo perduto pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra magazzino in base alla dichiarazione riepilogativa. Abbiamo implementato poi di 105 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale per indennizzi per riuscire a risarcire le imprese agricole danneggiate da gelate e brinate verificatesi nell'aprile del 2021. è l'ampliamento del tempo di applicazione di questa misura aggiungendo anche i mesi di maggio e giugno e aggiungendo le grandinate che, come avete potuto vedere in questi ultimi tempi, hanno devastato gran parte del nostro Paese. Lo stanziamento finale sarà di ben

nel nostro Paese. Abbiamo presentato un ordine del giorno per proporre una soluzione su questo tema importantissimo. È stato approvato - ringrazio la Commissione bilancio - questa mattina. L'estate 2021 è stata la peggiore dell'ultimo decennio per il ripetersi di 517 eventi estremi (nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, grandinate, ondate di calore e soprattutto siccità). Tale situazione nell'ultimo decennio ha determinato un periodo di perdite pari a 14 miliardi di euro. Per fronteggiare questo problema importante di accedere al Fondo di solidarietà nazionale delle imprese danneggiate. Ricordo anche che c'è una misura molto rilevante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede la possibilità di attingere a delle risorse per contenere l'acqua. Noi conteniamo solo l'11 per cento dell'acqua piovana o che arriva dai ghiacciai delle montagne. Anche qui, bisogna dare modo ai nostri consorzi, alle nostre associazioni - l'ANBI l'ha chiesto più volte a gran voce - di poter attuare delle misure in grado di portare avanti questi progetti con una tempistica più lunga di quella prevista attualmente, cioè il 23 settembre. Per aiutare l'agricoltura italiana, le misure da realizzare sono ancora molte, qualcosa è stato fatto e siamo qui per approvare questo provvedimento.

questa è la mattinata delle feste, siamo tutti entusiasti dell'obiettivo raggiunto: 44 miliardi di di nuovo debito da aggiungere agli altri 150 che abbiamo già maturato, siamo tutti felici grazie a tutto oggi porta all'approvazione anche al Senato di un provvedimento che se fosse stato affrontato con questa filosofia dal maggio dello scorso anno probabilmente avremmo avuto molti meno problemi.

che più volte noi di Forza Italia abbiamo rilevato come questione banale: bastava capire quali erano i bisogni delle imprese, che sono l'unica struttura

copertura non soltanto nel momento in cui stava maturando la questione, ma per metterle in condizioni di salvarsi e ristrutturarsi ed essere pronte domani quando "mamma Stato" non sarà più lì a pompare denaro nelle casse, sul territorio e anche agli enti locali. Questo è l'elemento sul quale dobbiamo ragionare. Forza Italia si è subito posta l'obiettivo di dare una visione e mi dispiace per i colleghi, ma il nostro è forse l'unico partito che ha presentato un pacchetto nutrito di proposte di visione per i prossimi dieci anni, a partire dalla riforma fiscale e dalla riforma del lavoro,

spesso di quelli che ci guardano da fuori per vedere di poter tornare ad investire nel nostro Paese e la prima cosa con la quale si sono scontrati è la questione della giustizia. Oggi è aperto un dibattito significativo

che non è esattamente quello che volevamo noi, ma quantomeno è sicuramente un passo in avanti per un ripristino di alcune situazioni, dal momento che in questi anni, non certo grazie ai nostri voti,

Abbiamo capito che siamo l'unico Paese al mondo che fa pagare stipendi per il 160 per cento alle imprese e ai dipendenti non tocca nemmeno la metà?

che ha disintegrato il lavoro, cancellato il tempo determinato, tolto la flessibilità, ucciso i *voucher* e messo in ginocchio il sistema delle imprese italiano, che abbiamo scoperto che per il 70 per cento è stagionale: evviva!

ma non vogliamo redditi di cittadinanza, assistenzialismo, nulla di tutto questo. Vogliamo un mercato libero e serio che metta al centro le imprese. Questa è la prospettiva di Forza Italia; speriamo lo capiate anche voi. Signor Presidente, Governo, colleghi,

che hanno necessità di sostegno. Evidentemente il poco tempo che ho a disposizione mi impedirebbe di affrontare il testo nella sua interezza, quindi mi limiterò ad approfondire alcuni articoli di mio interesse,

Questo è un problema che in Assemblea conosciamo bene - è stato affrontato più volte - ma che conoscono bene anche nel Paese. Alcuni erroneamente potrebbero pensare che si tratti di un problema limitato a un settore specifico, quello delle costruzioni, ma in realtà non è così. Se, infatti, pensiamo che il gas naturale ha quasi triplicato il suo prezzo negli ultimi mesi, è evidente che diventa un problema che va ad incidere sulla vita quotidiana di tutti. Non a caso, le bollette del gas sono aumentate del 15 per cento, ma dovrei dire solo del 15 perché grazie all'intervento di questo Governo si è riusciti a limitare l'onere a carico delle famiglie a una percentuale dieci volte inferiore a quella che invece è stata la percentuale di rivalutazione del prezzo della materia prima.

L'articolo 3, comma 1, nello specifico, prevede 100 milioni in più per i Comuni montani a favore dei comprensori sciistici. Sappiamo bene che quel settore ha sofferto moltissimo a causa del Covid. ha reso sostanzialmente impossibile lavorare anche solo per un giorno, quindi il colpo che hanno subito è molto duro, e quello è un tipo di turismo che, invece, potrebbe dare molto alle nostre realtà, anzitutto perché destagionalizzata il periodo, visto che la maggior parte dei turisti viene nel nostro Paese d'estate - questo già da solo sarebbe un elemento molto importante - ma spesso rappresenta la differenza tra la vita e la morte per quelle realtà montane. Quindi, prevedere un intervento a favore dei comprensori sciistici è stato sicuramente utile e opportuno. L'articolo 7-*ter* prevede il recupero, la riconversione e la valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali.

hanno per competenza la possibilità di intervenire sul 20 per cento del territorio nazionale. Quindi, tutto ciò che serve a valorizzare queste aree evidentemente non può che avere una ricaduta positiva sul resto del Paese. Propongo pertanto uno spunto di riflessione. Come dicevo prima, i nostri borghi potrebbero diventare un valore aggiunto per il Paese. Occorre, però, che questi vengano resi idonei non solo per un turismo che spesso è del tipo mordi e fuggi, giornaliero, ma anche per coloro che dovessero o volessero decidere di rendere la propria vita compatibile con uno stile di vita completamente diverso da quello che sarebbe possibile nelle nostre realtà cittadine.

È solo uno spunto, come dicevo prima. È bene che siano state previste già adesso delle misure, ma, a mio avviso, la lungimiranza che un Governo dovrebbe avere, dovrebbe portarlo a prevedere un ulteriore investimento importante a favore di quelle realtà, in considerazione del fatto che l'obiettivo di consumo zero di suolo, previsto dall'Unione europea per il 2050, potrebbe far sì che quell'edificato acquisti valore anche in un'ottica di di salvaguardia e tutela del nostro territorio, appunto perché si tratta molto spesso di aree già edificate, che necessitano solo di interventi infrastrutturali. Un'ulteriore possibilità per fare in modo che quelle realtà raggiungano l'autosufficienza economica sta evidentemente nel potenziare e valorizzare le piccole produzioni locali, che a livello europeo spesso vengono pregiudicate, ma che sono invece uno dei nostri valori aggiunti. Chiudo con il riferimento all'articolo 9, che prevede misure a favore dei terremotati.

Non è stato possibile prevedere degli emendamenti a questo articolo perché, come già detto da alcuni colleghi, la scadenza del decreto lo ha reso sostanzialmente impossibile. C'è già molto nel decreto, quindi sarebbe stato imperdonabile che venisse fatto scadere, però un intervento, secondo me, era necessario e per questo ho presentato un ordine del giorno. Sostanzialmente le attività produttive delle aree terremotate non ricevono un contributo per l'IVA: i privati sì, le attività produttive no perché, potendo recuperare l'IVA avrebbero un vantaggio

e ulteriormente penalizzata dal Covid, è chiaro che quell'onere, che in alcuni casi potrebbe superare le centinaia di migliaia di euro, per alcuni non è sostenibile. In una prima stesura dell'ordine del giorno addirittura chiedevo l'esonero dal pagamento dell'IVA. Le difficoltà che avremmo avuto per arrivare a quello mi hanno portato a rimodularlo e a chiedere una riduzione. Spero che il Governo possa

del Governo, colleghe e colleghi, tralascio le considerazioni politiche su un decreto che il nostro ramo del Parlamento, il Senato, esamina in soli due giorni. Mi concentrerò, invece, sulle considerazioni più puntuali sul provvedimento. Il decreto al nostro esame è dedicato ai temi del sostegno al reddito e al lavoro. A quest'ultimo sono dedicate anche diverse norme di tipo ordinamentale raccolte in un unico titolo. Buona parte dei 43 miliardi di euro previsti sono impegnati per sostenere le attività economiche e, al contempo, per sostenere la ripartenza di chi è motore di queste aziende oppure ci lavora. In sostanza, questo è ancora un provvedimento di urgenza, ma tendente ad uscire da un'emergenza, guardando alla ripartenza del Paese. Il valore di questo decreto è proprio nell'enorme iniezione di denaro che il Governo ha fornito complessivamente al sistema Italia, dando ossigeno a un'economia che in parte era entrata in terapia intensiva e che ora potrà uscirne in piedi. La conseguenza dei *lockdown* totali o parziali ha causato un rallentamento dell'economia, che ha avuto un effetto domino su tutta una serie di filiere e di settori tra loro collegati. C'è nel decreto, quindi, anche il tema del blocco parziale dei licenziamenti. Lo sblocco ha interessato aziende la cui attività è stata limitata dai *lockdown*, ma ha coinvolto anche tantissime altre aziende*.* Adesso, senza entrare nel merito delle differenti situazioni di crisi aziendali, una cosa va detta anche dalla mia parte politica. Non si può licenziare senza che ve ne siano le condizioni, senza preavviso e senza avere prima attivato gli ammortizzatori sociali a disposizione. Usciremo da questa emergenza e dobbiamo capire che servono disposizioni nuove che non lascino a casa i lavoratori, ma li ricollochino preparandoli ai nuovi lavori. Occorrono norme che premino la produttività, che incentivino l'innovazione e che quindi rendano più competitive tutte le nostre attività economiche. Inoltre, è fondamentale un sistema di ammortizzatori sociali che copra sia il lavoro dipendente che quello autonomo. Alla base di tutto è però necessaria anche una pubblica amministrazione più snella, più digitale, più efficiente, più colloquiante con i cittadini e le imprese. E va assecondato l'ottimo lavoro del ministro Brunetta in tal senso. Noi, nondimeno, riteniamo che dalle disposizioni di questo decreto si debba partire non per creare una nuova stratificazione normativa, ma per adottare una legislazione a regime, che sia anche resiliente per eventuali ulteriori situazioni di emergenza. Andando sul concreto: il reddito di cittadinanza è una misura di cui attendiamo una riforma, per destinare le risorse in parte ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali e in parte alla formazione continua dei lavoratori *(Applausi)*, tema per noi prioritario. Che il reddito di cittadinanza abbia funzionato solo in parte come misura di contrasto alla povertà lo dimostra il fatto che è servito anche un reddito di emergenza, che è pure rifinanziato in questo decreto. del lavoro (ANPAL) e i centri per l'impiego (CPI), al fine di destinarle realmente alle politiche attive, attraverso le imprese e le agenzie private di collocamento, che con le aziende dialogano quotidianamente e puntualmente. Alle tradizionali macrovoci di spesa pubblica che sono appunto i redditi pubblici per 174 miliardi, alle pensioni per 236 miliardi, si è aggiunta quella voce che ha raggiunto nel 2020 i 144 miliardi di oneri INPS per gli interventi sociali, che sono già a carico della fiscalità generale. Poiché con questo decreto siamo di fronte ad una vera e propria manovra economica, allora è necessario ragionare anche in termini di programmazione di bilancio. L'invito è quindi a lasciare le bandiere ideologiche che come abbiamo visto corrispondono solo ad un consenso temporaneo. È necessario ragionare in termini di riprogrammazione a lungo periodo pianificando quelle riforme del mercato del lavoro che lo rendano più dinamico e non più ingessato, come dicevano anche i colleghi di Forza Italia intervenuti prima di me. Ce lo hanno dimostrato le grandi economie, come quella americana, che è un esempio per tutti, dove il lavoro è ripartito con la ripartenza delle imprese. Al contempo preparando un sistema di ammortizzatori che sia predisposto, ma che venga attivato solo in caso di necessità. Questa pandemia e i tanti interventi normativi che l'hanno accompagnata ci hanno insegnato che l'essere cittadini e l'avere identità di esserlo ci viene dal possedere un lavoro vero ed equamente retribuito. la possibilità di cambiarlo, migliorando la propria preparazione professionale, si realizza con una reale strutturazione di una formazione continua per tutti, ma proprio tutti i lavoratori. definitiva, ripartiamo dai 42 articoli del titolo IV del provvedimento, dalle buone norme esistenti e, utilizzando al meglio le risorse del PNRR, realizziamo una riforma duratura e condivisa sui temi del lavoro e della previdenza. *(Applausi)*.

oggi in Aula discutiamo del decreto-legge sostegni-*bis*, un provvedimento che vale 40 miliardi, un provvedimento importante e molto atteso da aziende e lavoratori. Ne discutiamo oggi e domani verrà posta la fiducia. Certo, avrei voluto che il dibattito parlamentare di queste ultime settimane fosse incentrato sulla situazione attuale, sul benessere o sulle problematiche delle attività e sulla tenuta dei posti di lavoro. Invece qui in Senato, in queste ultime settimane, il lavoro è stato orientato su un disegno di legge che riguarda i temi importanti come i diritti civili, ma forse non così impellenti come la necessità di garantire a tutti, ribadisco a tutti, il primo e fondamentale diritto, il lavoro. Il provvedimento consta di 77 articoli con più commi e questo dà una fotografia su quanto il lavoro del Governo e della Camera in questo caso sia stato importante per riuscire a coprire tutti i comparti e settori colpiti dalla pandemia. Se facciamo una somma di tutte le risorse che lo Stato ha stanziato in questo ultimo anno e mezzo, ci rendiamo conto che, tra ristori e sostegni, le cifre erogate non si allontanano molto dall'importo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sappiamo bene che ristori e sostegni, come il differimento delle scadenze fiscali, non sono sufficienti a colmare le perdite subite dalle chiusure e quindi dal blocco delle attività produttive; sono esclusivamente dei palliativi, in attesa che la ripartenza riporti questa ruota, che si è bloccata, a girare meglio per tornare alla normalità o ad una pseudo normalità.

tenendo conto dell'effettivo calo di fatturato nel periodo pandemico, quindi da aprile 2020 a marzo 2021. Grazie alla Lega, la soglia di fatturato per le aziende è stata alzata da 10 a 15 milioni ed è stata prevista È stato ampliato di ulteriori 100 milioni il Fondo nazionale per la montagna, penalizzata per la mancata stagione invernale. Grazie al ministro Garavaglia, che ha portato la voce preoccupata e allarmata del settore, sono stati stanziati nei due decreti-legge sostegni 800 milioni. Sempre grazie alla Lega sono stati inseriti ulteriori 30 milioni destinati ai comprensori sciistici da destinare alla sicurezza e all'innovazione tecnologica di piste e impianti. è anche il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con una dotazione iniziale di 100 milioni, incrementata di ulteriori 40 milioni; positiva è anche la modifica relativa ai tempi di chiusura necessari per accedere ai fondi che, dai quattro mesi previsti inizialmente, si riduce a 100 giorni. è anche il contributo a fondo perduto di 77 milioni per piscine e palestre, solo per citare alcuni provvedimenti. Di certo la perdita della stagione invernale ha di fatto messo la parola fine su diverse attività. Questa mattina nei giornali viene data rilevanza alla notizia della vendita di ben cento alberghi in Trentino; alcune attività, infatti, erano già in difficoltà prima della pandemia, altre invece, stante le difficoltà, hanno alzato le mani e abbassato le serrande, un segnale forte e importante, ma soprattutto impattante per comunità piccole dove il turismo è il settore economico principale. Perdere un'attività economica non può essere relegato ad una mera perdita economica, perché di fatto lede l'equilibrio di una comunità: mi riferisco alla salvaguardia di tradizioni e cultura e, visto che provengo da una minoranza linguistica, anche alla perdita della stessa. Tutto questo per una mancanza di liquidità che porta anche i più convinti a cedere davanti all'inevitabile. In questi giorni la stagione turistica è partita e, se da parte dei nostri connazionali c'è grande voglia di raggiungere le località turistiche, gli albergatori, i ristoratori e gli esercenti si trovano ad affrontare un'altra difficoltà: la carenza di personale. Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l'economia del Paese: vale il 13 per cento del PIL, occupando il 7,1 per cento degli occupati. Il settore lamenta forti criticità a reperire forza lavoro: mancano tra i 150.000 e i 200.000 lavoratori, cioè un quarto della forza lavoro richiesta. Una delle motivazioni indicate è l'esistenza del reddito di cittadinanza che, per come è stato pensato e strutturato, presenta diverse criticità e, anche se nel momento pandemico è stato sicuramente uno strumento utile al sostentamento dei cittadini, ha di fatto dimostrato tutte le criticità

su un totale di 1.369.000 persone tenute alla sottoscrizione del patto di lavoro, solo 352.000 persone hanno avuto almeno un rapporto di lavoro, pari al 25,7 per cento sempre al 31 ottobre, però, i contratti di lavoro attivi erano solo 192.000, in quanto solo il 15,4 per cento dei beneficiari ha firmato un contratto a tempo indeterminato, mentre il 4,1 per cento ha avuto un contratto di apprendistato e il restante 65 per cento un contratto a termine. Questo sta a significare una inadeguatezza del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il compito del legislatore in questo caso è mettere in campo le modifiche necessarie, affinché le criticità emerse trovino soluzione, senza buttare su lavoratori o imprenditori sentenze di parte. Concludendo, Presidente, per il rilancio della nostra economia serve dare certezze per il futuro, garantendo continuità alle attività produttive che a loro volta generano lavoro. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio molto di aver sollecitato questo mio intervento in Assemblea su fatti che sono gravissimi. Ciò è necessario per darmi la possibilità di condividere con tutto il Parlamento una ricostruzione dell'accaduto, dell'accaduto, dei fatti, degli interventi dell'autorità giudiziaria e del Ministero e, soprattutto, di condividere alcune linee di intervento che stanno maturando, un po' più ad ampio spettro, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e presso il Ministero tutto, sui problemi del carcere, per aggredire le cause più profonde e più radicate che hanno permesso, o quantomeno non hanno impedito, fatti così gravi. La data oggi reca una coincidenza storica, che non possiamo non ricordare. È il 21 luglio e in questa stessa data di venti anni fa, esattamente a Genova, durante i giorni del G8, succedevano fatti di una violenza altrettanto inaudita. E allora è nostro dovere - oggi parleremo di Santa Maria Capua Vetere - riflettere sì anzitutto sulla contingenza, ma anche sulle cause profonde che hanno portato, un anno fa in quel carcere, a un uso così smisurato e insensato della forza. Fatti di questa portata richiedono una risposta immediata da parte dell'autorità giudiziaria, che deve far luce su tutto e accertare le responsabilità penali. Ma fatti di questa portata sono spie di qualche cosa che non va e che dobbiamo indagare. Dobbiamo intervenire con azioni di lungo periodo perché non accada mai più. Come ho già avuto modo di dire proprio lì a Santa Maria Capua Vetere, durante la visita con il Presidente del Consiglio, questi gravissimi fatti, oltre a sollecitare la nostra più ferma condanna, reclamano un'indagine più ampia, perché si conosca quanto successo in tutti gli istituti penitenziari nell'ultimo drammatico anno, un anno in cui la pandemia ha esasperato le condizioni del carcere, già difficili per il sovraffollamento, per la fatiscenza delle strutture, per la carenza del personale e per tante altre ragioni. E allora guardiamo in faccia a tutti i problemi, spesso cronici, dei nostri istituti penitenziari, affinché non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti, né contro gli agenti della Polizia penitenziaria, troppo spesso aggrediti, né contro tutto il resto del personale, che opera in condizioni difficili. Il carcere è specchio della nostra società ed è parte della nostra Repubblica; non possiamo rimuoverlo dallo sguardo e dalle nostre coscienze. Violenze e umiliazioni si sono viste a Santa Maria Capua Vetere; violenze e umiliazioni inflitte ai detenuti, che recano una ferita gravissima alla dignità della persona, alla persona di chi le ha subite, ma sono in spregio anche alla dignità di chi le ha commesse. La dignità è pietra angolare della nostra convivenza civile, come ci chiede la Costituzione, che è nata - ricordiamolo sempre - dalla storia di un popolo che ha conosciuto e pagato sulla sua pelle il disprezzo del valore della persona e per questo si pone a scudo di tutti, specie di chi si trova in posizione di maggiore vulnerabilità. L'uso della forza, anche da parte di chi legittimamente lo può esercitare, sia sempre strumento di difesa, di difesa soprattutto dei più deboli, mai di aggressione, mai di violenza, mai di sopruso. I fatti sono noti, sono tristemente noti, anche per il meritorio lavoro della stampa, che ringrazio, perché ha acceso davvero i riflettori su una vicenda che non poteva rimanere nascosta. Il 6 aprile dello scorso anno è stata disposta una perquisizione straordinaria nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse, che hanno coinvolto agenti della Polizia penitenziaria e personale dell'amministrazione, sono gravi. Esse riguardano delitti di concorso in torture pluriaggravate, maltrattamenti, lesioni personali, falso in atto pubblico, calunnia, favoreggiamento, frode processuale, depistaggio. Tutti i delitti sono pluriaggravati dalla minorata difesa, dall'aver agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, con abuso di potere, in violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica, con l'uso delle armi e per l'aver concorso negli eventi un numero di persone superiore alle cinque unità. Invero le notizie della stampa già dallo scorso autunno riferivano di violenze e indagini in atto all'interno di quell'istituto. C'era già stata un'interrogazione parlamentare in proposito. Mi sono chiesta e ho chiesto all'amministrazione penitenziaria come mai i fatti emersi non avessero dato luogo a un'azione da parte del Ministero. Mi è stato spiegato nelle ultime settimane - ed è stato confermato dall'autorità giudiziaria - che l'amministrazione penitenziaria aveva chiesto informazioni ai giudici che procedevano, ma il giudice procedente non poteva rispondere per ragioni di segreto investigativo. È per questo che - come spiegherò più avanti - tutte le iniziative di cui darò conto nell'ambito del Ministero sono successive ai fatti emersi alla luce della cronaca da parte dei giornali. Di quali fatti si tratti lo sappiamo. Non voglio insistere sulle immagini che tutti conosciamo, ma non posso togliermi dallo sguardo e dalla mente - ad esempio - l'immagine di un detenuto costretto a inginocchiarsi prima di essere colpito. non solo violenza, ma proprio il gusto dell'umiliazione. Un altro caso riguarda un detenuto in carrozzella. E tutto avveniva sotto le videocamere che hanno ripreso tutto.

Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, la perquisizione straordinaria del 6 aprile è stata disposta fuori dai casi consentiti dalla legge, non sono state rispettate le forme richieste e non vi è stato alcun provvedimento del direttore, che è l'unico che può disporre e ha il potere di farlo. Secondo quanto emerge dagli atti - cito dall'ordinanza - vi sarebbe stato solo un provvedimento orale, e cioè un ordine verbale, per svolgere una perquisizione a scopo dimostrativo, preventivo e satisfattivo, finalizzato a recuperare il controllo del carcere e appagare presunte aspettative del personale della Polizia penitenziaria. Queste le parole dell'ordinanza del gip. Il giorno prima c'era stata una rivolta in carcere e nella sua ordinanza il gip riporta alcune intercettazioni che - per esempio - parlano di un segnale per riprendersi l'istituto. In ogni caso, sempre dalla lettura degli atti, emerge che non era una perquisizione volta a ricercare strumenti atti all'offesa presuntivamente detenuti dai detenuti, o altri oggetti che non potevano essere tenuti in carcere, ma nella quasi totalità dei casi - leggo testualmente dal provvedimento - era mera copertura fittizia per la consumazione di condotte violente, contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse. Si tratta di contestazioni di una gravità inaudita. Ancora sui fatti, permettetemi di far riferimento alla situazione di un detenuto, di cui forse avete letto sui giornali.

Il gip scrive che non vi sono le evidenze che dimostrino che il detenuto sia morto in conseguenza dei colpi e delle ferite riportate il 6 aprile, ma soggiunge anche che è possibile che il sopravvenuto decesso sia da ricondurre all'assunzione di farmaci resi necessari per curare quelle ferite e contusioni, che, sommati ai farmaci che assumeva per la sua malattia (la schizofrenia), hanno provocato un arresto cardiaco. Mi è stato chiesto - e ripeto qui - cosa ci faceva un malato di schizofrenia in carcere. E questo apre un altro capitolo, un'altra riflessione, anch'essa resa ancora più drammatica ed esasperata dopo l'anno di pandemia: la tutela e la cura della salute mentale dentro e fuori dal carcere. *(Applausi)*. Abbiamo davvero strutture necessarie? Questo punto meriterà un grande approfondimento. Tra l'altro, la Corte costituzionale ha chiesto al Ministero della giustizia, alle Regioni e al Ministero della salute dati e approfondimenti per un'istruttoria che sta conducendo. Non possiamo lasciare le cose così come sono; sono stati fatti passi molto importanti con la chiusura degli OPG, ma attualmente le attività di cura e di supporto ai malati sono altamente insufficienti. Torniamo al nostro caso. Che cosa è successo dopo che l'autorità giudiziaria ha reso note una serie di misure cautelari che sono state prese nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria e anche di personale dell'amministrazione? Vi risparmio la lettura dei provvedimenti per dei provvedimenti per pura ragione di tempo; non li leggo analiticamente, ma chiedo sin da subito alla Presidente se posso consegnarli, in modo tale che in totale trasparenza ci sia l'analitica descrizione di tutti i provvedimenti assunti. Posso dire sinteticamente che tutte le unità di personale penitenziario che sono state raggiunte da una misura cautelare sono state anche immediatamente sospese dal servizio. È stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio per otto mesi anche il provveditore regionale della Campania, e alcune ulteriori misure di sospensione dal servizio hanno riguardato altre persone indagate pur non coinvolte dai provvedimenti di sospensione cautelare (una sospensione che è nella facoltà del Ministero decidere di assumere). Analogamente, sono stati sospesi il direttore reggente *pro tempore* del carcere e il vice direttore. Preciso che l'attuale direttrice non era presente il giorno dei fatti, perché assente per malattia, e non è indagata. Di queste misure cautelari, alcune sono anche state revocate per vari motivi: in particolare, una per un errore di identificazione dell'indagato, e un'altra perché il gip ha ritenuto non necessario proseguire con la misura cautelare. In breve, il totale complessivo delle unità di personale dell'amministrazione sospese a vario titolo è di Rimangono altri indagati per i quali il gip ha specificato che non v'è certezza della loro presenza e per questo ha respinto la richiesta di misura cautelare. Ovviamente, su questo punto si attendono gli sviluppi dell'indagine prima di ogni altra valutazione. Per quanto riguarda i detenuti, tutti coloro che sono stati coinvolti sono stati trasferiti, come si fa normalmente per ragioni anche di sicurezza in altre sedi, dentro o fuori dal territorio.

alla contestazione di questi fatti, quando abbiamo ricevuto il provvedimento dell'autorità giudiziaria e quando sono emerse le immagini sui giornali,

dei detenuti. L'esigenza era innanzitutto capire come fosse stato possibile e quali fossero le informazioni a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; chiedere di allargare la prospettiva, perché - lo sappiamo tutti - in molte carceri italiane ci sono state tensioni che hanno messo in grande agitazione il carcere, sia per le aggressioni che hanno riguardato il personale, sia per il contrario, sia per riflettere un po' sulle cause più profonde. Se sono successi fatti come quelli di cui stiamo parlando in quest'Aula, è perché troppe cose non hanno funzionato, e non da ieri, non da un anno fa, ma da un tempo più lungo. Quello che è accaduto a Santa Maria di Capua Vetere - lo ha detto il presidente Draghi durante la visita - è una sconfitta per tutti noi. Le responsabilità penali sono individuali e personali. Non si vuole lenire nulla da questo punto di vista, non ci sono giustificazioni o attenuanti, ma noi non avvertiamo la responsabilità del contesto in cui è stato vissuto il carcere, soprattutto nell'ultimo anno? Io ho voluto approfondire personalmente, sentendo i rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria, e ho voluto confrontarmi con tutti i provveditori, che sono le articolazioni territoriali dell'amministrazione penitenziaria sul territorio. È stata disposta una commissione ispettiva interna, in modo tale che la stessa amministrazione possa andare anche prima, anche indipendentemente dall'attività giudiziaria, a ricostruire problemi problemi e situazioni di tensione, soprattutto in riferimento a quelle realtà in cui già sappiamo esservi delle spie di tensioni avvenute nell'ultimo anno. La commissione visiterà tutti gli istituti penitenziari interessati da manifestazioni di protesta, denunce o segnalazioni inerenti ai gravi eventi occorsi dal marzo del 2020. Occorre approfondire la dinamica, verificare la legittimità e la correttezza di ogni iniziativa adottata. Credo che sia davvero importante che, soprattutto in un'amministrazione chiusa come l'amministrazione penitenziaria, il Ministero nelle sue articolazioni sappia indagare al suo interno. Deve capire e portare alla luce le eventuali violazioni e criticità. Credo che su questo punto qualcosa sia mancato, che ci sia stata una mancanza da parte del Dipartimento dell'amministrazione ministeriale, almeno in questa occasione. Occorre indagare sugli episodi critici, ma anche andare alla ricerca delle cause più profonde e, soprattutto, creare condizioni materiali e normative per evitare ogni ulteriore nuova violenza. Il confronto con la polizia, con l'amministrazione, con i provveditori, con i vertici del DAP mi ha dato molti spunti di riflessione: ad esempio, mi segnalavano che molti degli agenti coinvolti in questa brutta vicenda era personale della Polizia penitenziaria normalmente non più adibito alla sorveglianza, ma preposto ad altre funzioni; mi hanno sottolineato l'età avanzata di molti di loro e in generale un innalzamento dell'età media di tutti gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, anche per le difficoltà del *turnover* e dell'assunzione di nuovo personale. Tutti mi hanno ribadito la fortissima tensione che in quei mesi di pandemia si viveva negli istituti penitenziari. Bisogna capire e cogliere tutto questo, capire e agire. Oltre a ciò che vi ho detto al riguardo della salute mentale, ho individuato almeno tre linee di priorità che debbono impegnare il Ministero sin da subito:

è un problema enorme, e non solo per il sovraffollamento negli spazi, ma anche per il degrado di moltissimi ambienti. Mettere piede in un carcere - come di nuovo mi è capitato di fare, per esempio a Santa Maria di Capua Vetere - è istruttivo. Non mi stanco mai di ripetere una frase che ha segnato profondamente il mio sguardo verso quel mondo, che è quella di Piero Calamandrei, quando inizia, sul carcere, dicendo: «Bisogna aver visto». È difficile descrivere le condizioni ma, una volta che si sono viste le immagini, si conficcano nella memoria. I tanti di voi che hanno visitato le carceri italiane lo sanno. Ho in mente le immagini di tutti i detenuti attaccati alle grate che cercavano di salutare il Presidente; la vista di un istituto che ribolliva per il calore, la fatica a respirare in determinate celle; la notizia che non conoscevo che in quel carcere non c'è l'acqua corrente, perché è stato progettato senza pensare agli allacciamenti necessari e, quindi, l'acqua arriva ai detenuti nelle taniche ogni giorno. Possiamo pensare che un ambiente così degradato sia favorevole allo scopo che il carcere ha? Possiamo parlare di rieducazione quando le strutture sono in queste condizioni? Possiamo immaginare le condizioni di lavoro di un mestiere difficilissimo che viene compiuto da chi svolge le più varie funzioni dentro il carcere (la Polizia, l'amministrazione, gli educatori,

Occorre rimodernare e aggiustare ciò che c'è, ma anche ampliare per il problema del sovraffollamento. Sapete che con i fondi del PNRR è stata prevista la costruzione di di otto nuovi padiglioni. Ci tengo a ribadirlo perché ho chiesto alla commissione dell'architettura penitenziaria che sta lavorando su questo di ampliare non solo i posti letto, pur necessari, ma anche gli spazi di socialità.

che quei fatti potessero emergere alla luce dei nostri occhi proprio in virtù della videosorveglianza, che è qualcosa che chiedono tutti: lo chiedono i detenuti e lo chiedono gli agenti. È, infatti, a tutela di tutti. *(Applausi)*. Le aggressioni colpiscono Le aggressioni colpiscono il personale che lavora e colpiscono i detenuti. Quando c'è tensione, nessuno esce vittorioso. Poi occorre intervenire in modo significativo sulla dotazione del personale. Ci sono carenze gravissime in tutti gli organici (la Polizia, gli educatori, il personale dell'esecuzione penale esterna). Abbiamo ripreso i concorsi che erano bloccati per la pandemia; si stanno concludendo, ma moltissime carceri italiane non hanno un direttore,

Ancora ci sono i problemi delle donne con i figli in carcere. Potete immaginare strutture così che non hanno un punto di coordinamento, un vertice ultimo e sottoposti a continue criticità? Permettetemi un ultimo punto che mi sta particolarmente a cuore anche perché, di nuovo, è una riflessione frutto dell'ascolto dei protagonisti. Il personale della Polizia, il personale dell'amministrazione e tutti gli educatori chiedono non non solo una formazione iniziale (lo studio che serve per superare il concorso e che magari dà un'istruzione su come muovere i primi passi dentro realtà così complesse), ma una formazione permanente che nutra la cultura di cosa vuol dire rieducare dentro un carcere e che dia anche indicazioni operative su come misurare, quando è necessario - per esempio - l'uso della forza, come reagire di fronte alle più varie situazioni di crisi. *(Applausi)*.

per ricordare il titolo di un famoso libero di Foucault - non è solo sorvegliare e punire, ma è anche accompagnare nel percorso di rieducazione tutti i detenuti garantendo ordine e sicurezza e partecipando a un lavoro essenziale non solo per tutte le persone che vivono dentro il carcere, ma per tutta la società, perché chi vive in modo costruttivo il periodo della pena della reclusione è anche una persona meno incline alla recidiva. Non dimentichiamo questo aspetto. È anche per ragioni di sicurezza generale che dobbiamo conformare sempre di più il tempo della pena a quello che la Costituzione ci richiede: che la pena sia rieducativa. *(Applausi)*. Anche per questo abbiamo avviato un gruppo di lavoro presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per riflettere su cosa è stata la formazione fino adesso e che cosa deve diventare, diventare, lungo linee direttrici che nutrano la cultura ma diano anche indicazioni pratiche. I fatti di Santa Maria Maria Capua Vetere hanno squarciato un velo, forse in un modo un po' drammatico e violento, ma adesso la realtà del carcere italiano è davanti agli occhi di tutti, davanti agli occhi del Governo, che ha visto, anche con la visita in prima persona del Presidente del Consiglio, un fatto che non è passato inosservato in tutta la realtà carceraria. La visita del Governo, oltre ad essere un fatto simbolico anche di vicinanza e di presenza laddove c'è stata una ferita così grande, è anche un'assunzione di responsabilità. Il Presidente del Consiglio ha concluso quella sua visita dicendo che il Governo sa e non vuole dimenticare. Per non dimenticare, bisogna cominciare subito un'azione anche concreta di miglioramento e di risanamento di problemi endemici delle carceri italiane. *(Applausi)*.

abbiamo sentito dalle sue parole la ricostruzione di quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere e i provvedimenti che intende prendere il Governo per ricucire la ferita nello Stato di diritto che il pestaggio, giuridicamente qualificato come tortura, e i tentativi di depistaggio successivi hanno inferto nell'opinione pubblica, nella coscienza collettiva o almeno in quella parte - spero vasta - che considera anche i detenuti soggetti di diritto. So che lei ha a cuore questo tema e lo ha dimostrato da Presidente, portando la Corte costituzionale nelle carceri. Non è inutile da parte mia, in premessa, ribadire l'importanza del corpo di polizia penitenziaria nella gestione di un mondo complesso e difficile come quello delle carceri. Lo ha detto anche lei: strutture spesso fatiscenti, sovraffollamento, carenza di personale, di direttori, di educatori, psicologi, mediatori culturali. Proprio per queste motivazioni, al ringraziamento per tutti coloro che si adoperano con coscienza e dedizione, che ho potuto apprezzare nelle mie precedenti funzioni di magistrato, non può non corrispondere la più ferma e determinata condanna per quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere e temo - magari in forme meno gravi, ma comunque sempre inaccettabili - in altri istituti. Le immagini, lo scambio di messaggi tra gli indagati denunciano non un momento di follia - l'ha detto lei: una fredda azione - ma un sistema collaudato di violenza con un suo nome in codice, la complicità e la connivenza di funzionari di ogni ordine e grado, la consapevolezza della gravità dei fatti, il tentativo di cancellare le tracce, la determinazione nel depistare le indagini, la rabbia nel non esserci riusciti. Com'è possibile che, a seguito in tutto ciò, il DAP e il Ministero non siano intervenuti per più di un anno? Lo ha chiesto anche lei. Come è possibile che i principali responsabili siano rimasti al loro posto per tutto questo tempo? Gli avvisi di garanzia dell'11 giugno 2020 avrebbero dovuto consigliare in via cautelativa almeno il trasferimento degli indagati, che così hanno avuto la possibilità di fare pressione sui detenuti e indirettamente sui loro familiari per ritirare le denunce. Come si può far stare vittime e carnefici a convivere nella stessa comunità? E aggiungo il paradosso che ora a pagare le conseguenze dei pestaggi siano gli stessi detenuti, alcuni dei quali trasferiti a centinaia di chilometri dalle loro famiglie, non certamente i camorristi detenuti che sono rimasti fuori da tutto questo. Dispiace, al di là del cambio di Governo e del Ministro, che nulla sia accaduto prima dell'intervento della magistratura. Avremmo tutti preferito che fossero l'amministrazione penitenziaria e il Ministero a muoversi in anticipo, in autonomia, sulla scorta delle particolareggiate denunce del Garante dei detenuti della Campania, e non con una gestione burocratica di relazioni - evidentemente non corrispondenti alla realtà, viste le imputazioni di falso - che hanno portato il suo predecessore a parlare di una doverosa azione di ripristino della legalità. Per il rispetto che abbiamo della legge, per l'amore che nutriamo verso i principi costituzionali, non possiamo derubricare tutto questo a un episodio. Non possiamo cavarcela con la retorica delle mele marce. Siamo ancora in tempo per intervenire con forza. Le chiediamo di prendere al più presto i provvedimenti annunciati, come previsto dalle norme, e nel contempo di accelerare i concorsi, aumentare il numero degli agenti di Polizia penitenziaria e degli altri operatori e di migliorarne la formazione. Sappiamo che sono molti i problemi delle nostre carceri, e li ho elencati in premessa; abbiamo il dovere di intervenire per risolverli, per ripensare completamente il sistema carcerario da tutti i punti di vista - come ha giustamente sottolineato lei - l'intera architettura carceraria, a partire dalle funzioni, che vanno certamente contemperate, di sicurezza sociale e rieducazione. Non possiamo accettare che chi è chiamato a mantenere l'ordine e a garantire la correttezza della vita degli istituti

con tempi supplementari e questo aveva dato adito a varie contestazioni. Lo abbiamo stabilito e quindi, la pregherei di rispettare le regole come le rispettano tutti.

Grazie anche perché, di fronte a fatti gravissimi come quelli di cui abbiamo sentito

la forza con la quale si è sostenuta quell'iniziativa siano una cosa importante, perché credo che dimostrino la volontà del Governo, del Parlamento e delle istituzioni di fare piena luce e fare giustizia su quello che è successo. Signora Ministra, vogliamo fare piena luce su quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere, ma anche su altre vicende che sono aperte e penso ai 13 morti che ci sono stati durante le rivolte, su cui serve chiarezza. Ritengo che questa iniziativa, l'aver acceso con tanta forza questo faro, possa e debba essere anche un'occasione per un sussulto, per mettere mano in fretta e concretamente alla situazione delle carceri. Certo, dobbiamo impostare riforme più complessive, ma credo che servano anche misure da mettere in campo Il Parlamento deve fare la sua parte. Abbiamo chiesto e proposto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta proprio sulle violenze nelle carceri,

aumentate le aggressioni agli agenti e agli stessi operatori. C'è un clima di violenza all'interno delle carceri le cui ragioni vanno indagate, non basta giustificarle con la sovrappopolazione. Sicuramente c'è un problema di spazi trattamentali insufficienti, per cui va benissimo che nel PNRR si sia stabilito di finanziare non solo più posti, ma soprattutto più spazi trattamentali. Certamente hanno pesato il Covid, come ha detto anche lei, signora

che cosa dobbiamo tenere dei momenti di comunicazione con l'esterno che si sono creati durante Dobbiamo sapere - l'ha detto lei, signora Ministra, e l'ha detto bene - che c'è bisogno che il territorio e le istituzioni si occupino del carcere

controllo e prevenzione. Pesano poi certamente le condizioni di lavoro difficili in cui si sono trovati spesso a operare i lavoratori. Ministra, voglio dire solo una cosa. Come si riparte dopo il Covid? Credo che dobbiamo fare questa riflessione adesso; bisogna riaprire le attività,

lo stato di emergenza, signora Ministra, servirà anche prorogare le misure che hanno funzionato e che abbiamo inserito per ridurre il sovraffollamento nelle carceri. *(Applausi)*.

citando Calamandrei, Foucault e l'articolo 27 della Costituzione, e andando altresì a confermare una cultura della giustizia riparativa

è importante, se vogliamo essere considerati una società civile, che si prende cura degli errori che la società stessa mette in atto.

c'erano indagini già in corso e quindi non è stato possibile rispondere sui fatti specifici di Santa Maria Capua Vetere. Purtroppo però avevo già avuto modo di presentare a marzo un'altra interrogazione sui fatti accaduti a Modena e a Pavia e sulle agitazioni che riguardavano le carceri di Salerno, Napoli, Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari e Foggia.

nel marzo 2020 dalla situazione della pandemia. Quando tutti ricevevamo indicazioni sul distanziamento, sull'igiene e sulla cura, nelle carceri il sovraffollamento e la mancanza di sicurezza

erano stati preceduti da una rivolta. Cosa chiedeva quella rivolta, anzi, quell'agitazione, perché è stato è stato chiarito che non si trattava di una vera e propria rivolta, ma di un'agitazione? Sicurezza sanitaria,

ha parlato di costruire nuove carceri. Anche se la questione è chiaramente brutale, nel costruire nuove carceri,

per poter affermare i principi della Costituzione, occorre che le carceri siano vivibili *(Applausi)* e che vi sia uno spazio fondamentale per ciascun individuo.

Ho visitato circa 43 carceri del nostro Paese. Quello che ha descritto esiste in maniera abbastanza variegata nelle varie Regioni. Le porto l'esempio della Liguria,

capacità di garantire sanzioni necessarie e adeguate agli accertamenti di responsabilità individuali, perché solo di quello possiamo ragionare. Allo stesso tempo, però, spetta a noi, al Parlamento, darle un contributo, nel senso di realizzare le misure di prevenzione necessarie perché questi fatti non avvengano. Bisogna creare capacità di dialogo all'interno delle strutture carcerarie, tra detenuti e polizia penitenziaria. Sa meglio di me che oggi stiamo ragionando di un episodio molto grave commesso da alcuni uomini della polizia penitenziaria; non dimentico però - e lo sa meglio di me - che circa 400 poliziotti all'anno

che ciascuno si assuma la propria responsabilità e abbia cognizione dei diritti. Il diritto però significa anche sapere che, se si sbaglia, si

alle aspettative cui ho fatto riferimento, essenzialmente per garantire, attraverso misure di prevenzione, un clima diverso. Occorre il dialogo e la capacità di...

Mi spiace che ciò avvenga solo per fatti spiacevoli e non per le centinaia di segnalazioni consegnate proprio da quel mondo alle istituzioni. Purtroppo, però, spesso la politica non va nella direzione del buon senso e lo dico a malincuore,

e magari oggi quei video assurdi, che tutti abbiamo visto e commentato mesi fa, che hanno riempito i giornali e i telegiornali per settimane, non ci sarebbero neppure stati. Invece eccoci qui oggi a discuterne. Ognuno - per carità - farà la sua parte, avrà la sua teoria da mettere in campo, ci dirà più o meno le sue ricette e la giornata politica del mercoledì parlamentare finirà a commentare l'ennesima informativa letta in Aula dal Ministro. Questa è la prassi. Per carità, è legittimo, fa parte del nostro lavoro. Ma ci rendiamo conto che siamo qui a parlarne non perché il problema c'è, ma perché è successo l'ennesimo episodio spiacevole, sbagliato e da condannare? Per carità di Dio, non voglio giustificare nessuno: chi ha sbagliato pagherà. Ancora una volta, non siamo in grado di anticipare i problemi, ma dobbiamo rincorrere l'ennesimo disastro. *(Applausi)*. Signor Ministro, non entro nel merito di cosa sia successo, che ci ha spiegato benissimo; lo farà chi di dovere, non certo io oggi. Tuttavia, sui fatti di Santa Maria Capua Vetere mi limito a osservare che non credo sia da Paese civile vedere nomi e cognomi di poliziotti sbattuti sui giornali, ancor meno prima di un processo serio. Ritornando al ragionamento iniziale, al quale tengo molto, voglio ribadire a chiare lettere che stiamo dando un messaggio sbagliato. Infatti, dietro la nostra retorica parlamentare - l'ha sottolineato anche lei oggi si nasconde un messaggio di rassegnazione del Parlamento nel non voler affrontare questo tema nella sua totalità, che inizia proprio da quel campanello d'allarme che le sigle sindacali della Polizia penitenziaria più volte hanno espresso; basterebbe ascoltarle un po' più spesso. Caro Presidente, caro Ministro, cari colleghi, non siamo qui a parlare perché vogliamo porre rimedio a tutte le falle che negli anni hanno reso impossibile gestire il sistema carcerario. Non siamo qui a parlarne perché abbiamo colto, dopo esserci confrontati con chi svolge questo servizio sul campo, i problemi e il disagio quotidiano nel far andare avanti proprio la quotidianità all'interno di queste strutture. Parliamo di situazioni che vanno oltre il limite umano di sicurezza sul lavoro degli operatori stessi. In media, abbiamo un agente attivo ogni 70 detenuti, in alcuni casi ogni 100. Parliamo di un alto numero di detenuti psichiatrici e autolesionisti, che necessitano di cure diverse dagli altri. Oggi tutte queste tipologie sono rinchiuse e ammassate negli stessi istituti di detenzione e quasi sempre sono seguite dalla Polizia penitenziaria e non da persone formate per seguire questo tipo specifico di patologie più complesse. In proposito, farei una riflessione sulle falle della legge Basaglia, perché ne perché ne scaturisce un disagio che va a discapito della sicurezza degli operatori e dei detenuti stessi. *(Applausi)*. Non si può più far finta di niente. C'è un dato allarmante e crescente, di cui nessuno parla, che ha visto gli agenti di Polizia penitenziaria togliersi la vita per quella che in psicologia viene definita sindrome da *burnout*, un grave problema per gli agenti che oggi lavorano negli istituti di detenzione. Non solo: parlando di Polizia penitenziaria, scopriamo che mancano divise idonee e protezioni di difesa adeguate, così come, in generale, dovrebbero essere riviste altre dotazioni. Potrei continuare per ore a mettere sul tavolo problematiche per cercare di parlarne, ma in questo caso più che contenuti sul tavolo servono risposte immediate e urgenti. Gli agenti di Polizia penitenziaria sono persone, ragazzi e ragazze che si arruolano con la speranza di migliorare la loro vita, mettendosi a disposizione del prossimo. Non lasciamoli soli e non facciamo di tutta l'erba un fascio, di fronte a un episodio spiacevole e ingiustificato, ma entriamo seriamente nell'ottica di sistemare il sistema di detenzione italiano, proprio per evitare che queste situazioni avvengano ancora.

I fatti di Santa Maria Capua Vetere sono abominevoli e certamente non possono essere giustificati, soprattutto nei confronti di soggetti vulnerabili e considerando che a compiere questo tipo di violenze sono coloro che rappresentano lo Stato. Questi comportamenti offendono non solo gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria, ma tutti gli operatori penitenziari, che con mille difficoltà, quotidianamente, cercano di far funzionare gli istituti penitenziari, con scarsità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Sono molto preoccupata, perché constato il fallimento dello Stato. Lo dico con il cuore in mano, perché, prima di fare il politico, sono un tecnico. Ho dedicato tutta la mia vita professionale e privata alla legalità.

che con caparbietà cercano di portare avanti i percorsi di inclusione e di legalità, certamente la rieducazione e la risocializzazione previste dalla Costituzione diventano un'attività ardua. Teniamo infatti presente che la Costituzione parla di rieducazione e quindi il carcere interviene laddove la società, con la scuola e la famiglia, ha fallito e l'opera di rieducazione è certamente molto più complessa.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 carceri, nel corso degli anni, è stata una realtà scomoda. È stato più semplice adottare indulti, amnistie e provvedimenti ma in realtà non abbiamo affrontato il problema reale della necessità di adeguamento degli organici e degli spazi. Abbiamo avuto condanne da parte dell'Europa. Parliamo di educazione, ma l'Europa ci ha segnalato dove gli spazi sono ridotti e dove c'è una scarsa illuminazione e non dimentichiamo che ci sono ancora celle con il bagno a vista.

però, occorre visitare le carceri e andare nelle celle, ma non con visite preordinate. *(Applausi)*. Verifichiamo che in una cella di 21 metri quadrati ci sono sette detenuti, perché molto spesso i dirigenti penitenziari e i direttori,

stazionino negli istituti. Mi auguro che si metta mano a questa norma e che la si applichi. Non servono nuove leggi, ma la concretizzazione di quelle esistenti, in quest'attività di collaborazione con tutte le istituzioni. *(Applausi)*.

ha dimostrato che veramente stiamo affrontando un cambio di passo su questa materia, come più volte avevamo richiesto, rimanendo tuttavia inascoltati. Le sue parole su quello che è accaduto sono effettivamente confortanti e danno il segnale del suo impegno e soprattutto del rispetto di quello che ha assunto fin dal primo incontro con noi, quando ci ha detto che per lei il faro è la Costituzione.

non solo per quel che è accaduto durante l'anno della pandemia (e lei, in maniera assolutamente esaustiva, ha ricordato quegli accadimenti), che anche in precedenza avevamo avuto segnali del poco interesse nei confronti di quel settore. Basti pensare al fatto che la riforma Orlando necessitava dei decreti attuativi,

Finalmente ho sentito da lei parlare di giustizia riparativa e finalmente se n'è sentito parlare di nuovo, dopo tre anni, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, perché quello che è mancato fino a oggi è l'attenzione verso quel mondo. Di questo non possiamo

Le violenze all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno messo in crisi l'intero assetto sociale di uno Stato di diritto e segnalano lo sfasamento della collettività verso quella parte della della cittadinanza. È stato ben detto che finalmente anche i carcerati vengono trattati come normali cittadini e voi - lei assieme al presidente Draghi - ne avete dato ottima dimostrazione. C'è tanto da fare, C'è tanto da fare, però, perché dobbiamo prendere atto della situazione e del disinteresse manifestato soprattutto negli ultimi anni. Vogliamo

bene oggi, ancora una volta: con una buona educazione, si può avviare un percorso di reinserimento secondo i principi dettati dalla Costituzione, che purtroppo troppo spesso vengono dimenticati e messi da parte.

Questo è un clima che si viene a creare proprio a causa delle condizioni di disagio. Il problema del sovraffollamento delle carceri è ormai annoso ed era stato affrontato in maniera adeguatissima la scorsa legislatura,

Si è sempre fatto ricorso alla pena detentiva come unica risposta alla commissione di un reato per rincorrere demagogicamente il principio della certezza della pena.

avviarsi verso un percorso di vita nuovo e consono alle regole del diritto. Questa dignità spesso viene negata. È stato ricordato anche in precedenza che si vive spesso in condizioni di

badare al numero degli agenti di Polizia penitenziaria. Il suo annuncio sull'ampliamento della pianta organica sarà un fatto estremamente importante, così così come gli istituti che consentiranno l'utilizzo di pene alternative alla detenzione. La smetteremo quindi di rincorrere l'utilizzo della carcerazione come primo...

il degrado sono un fattore ormai comune da molti, troppi anni, in questo Paese in cui la politica ha pensato a fare altro. A volte, si sono costruiti anche penitenziari, ma sono stati lasciati come cattedrali nel deserto, senza essere stati nemmeno aperti.

il nostro apprezzamento, la nostra vicinanza e la nostra gratitudine ai 40.000 agenti, donne e uomini, della Polizia penitenziaria che tutti i giorni rappresentano lo Stato nei nostri penitenziari

Santa Maria Capua Vetere qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi, perché quello che si è visto non è accettabile, ma bisogna anche prendere le distanze da tutta una canea che abbiamo visto in questi mesi e giorni, in cui si è accusata la Polizia penitenziaria,

I nostri uomini in divisa nelle carceri non hanno a che fare con gli studenti della Bocconi, sia chiaro. Qui si parla di conoscere il carcere. Io conosco bene il carcere, lo conosco molto bene da tanti anni e conosco bene anche il personale che c'è lì dentro, quello in divisa e quello senza divisa, e anche gli utenti che frequentano i nostri penitenziari, quelli che in parte dobbiamo cercare di redimere, di portare sulla retta via, costruendo un percorso che possa reintegrarli nella nostra società. Purtroppo, sappiamo benissimo che lì dentro ci sono sacche larghissime di persone che commettevano reati gravissimi fuori e li continuano a commettere lì dentro. Francamente, rispetto alla soluzione che qualcuno ha proposto di di concedere pene alternative e di farli uscire dal carcere, bisogna vedere a chi e per quale motivo, altrimenti poi non possiamo venire qua in Parlamento o in televisione, con la lacrima sul viso, a dire che una tale donna è stata aggredita perché il tale, uscendo dal carcere in permesso, è andato lì e l'ha fatta fuori, l'ha uccisa, l'ha violentata, le ha fatto del male o le ha dato fuoco. Dopo è troppo facile fare il pianto del coccodrillo. Queste cose vanno prevenute. Ci sono personalità malavitose all'interno del carcere che non devono uscire fuori, ma devono stare dentro e scontare la pena. Signor Ministro, uno dei fattori che porta alla redenzione e al recupero dei nostri detenuti in carcere è il rispetto delle regole: nel carcere ci sono delle regole, non può vigere la situazione in cui lì dentro ormai abbiamo percorsi di vigilanza attenuata, per cui i detenuti sono liberi di fare quello che vogliono, spesso ovviamente offendendo. Questo non fa parte dei 1.234 casi di aggressione nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria;

è bene che chi si comporta in un certo modo nel carcere non debba avere sconti o facilitazioni di pena, anche per quanto riguarda la legge Gozzini. Non è accettabile che uno lì dentro si comporti così,

interessante sapere, anche nei confronti della magistratura, quanti di coloro che hanno commesso quei reati dentro i penitenziari, quelli che hanno spaccato tutto e sfasciato il carcere, hanno aggredito gli agenti nelle rivolte che ci sono state, abbia pagato in qualche modo per quello che ha fatto, in termini finanziari

un concorso fatto nel 2019, che riguardava 745 allievi agenti della Polizia penitenziaria, che è fermo da due anni. Questi ragazzi hanno passato l'orale e devono fare devono fare le prove attitudinali ed è due anni che aspettano di farle, perché non vengono assunti. Le volevo dire, Ministro, ma lei lo saprà meglio di me, che nei prossimi cinque anni ci saranno 12.000 agenti di polizia penitenziaria in meno, perché andranno in pensione, oppure saranno riformati. Bisogna cominciare a parlarne e a pensare adesso a quello che sta accadendo, perché già sono pochi adesso nei nostri penitenziari, nei prossimi anni saranno ancora meno. Un intervento su questo va fatto. Volendo metterla in positivo, Ministro, il fattore importante anche del suo presentarsi qui, alla Camera prima e al Senato adesso, a parlare di questi problemi è che voi volete vedere cosa sta succedendo e ve ne state rendendo conto. Certo che non possiamo dare la colpa a lei per quello che è avvenuto negli ultimi decenni, in cui una certa politica se n'è fregata di quello che avveniva nel mondo del carcere e ha preferito dare indulti, sconti di pena svuota carceri. Questo è stato fatto ovviamente colpendo anche i cittadini che poi hanno subito il reato e hanno visto, semmai, coloro che hanno commesso il reato uscire facilmente dal carcere o stare in giro a commettere altri reati. Sarebbe molto facile prendere da rispondere a ciò che l'Europa ci dice o ci impone, però noi dobbiamo fare ben altro e lei, Ministro, penso che in questo caso si sia resa conto di ciò che serve. Sono convinto che anche da parte di Fratelli d'Italia - noi siamo all'opposizione di questo Governo - se lei lavorerà nella direzione di affrontare i problemi e intervenire sulle realtà del mondo carcerario, troverà, come al solito, non un'opposizione fino a se stessa, ma un'opposizione propositiva e ovviamente troverà il nostro appoggio perché vogliamo la risoluzione dei problemi e non la polemica fine a se stessa. *(Applausi)*.

chiare, ma soprattutto pesanti e inequivoche. Lei ha toccato un argomento scomodo per la politica e su questa scomodità vorrei tornare. Direi che nella sua chiarezza c'è qualcosa di molto di più che identificare fatti spiacevoli avvenuti non solo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; c'è in ballo l'articolo 13 della Costituzione - è stato ricordato da molti - che esordisce dicendo che «la libertà personale è inviolabile» e dice anche che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Sul tema della libertà, sancita dall'articolo 13, è dall'inizio di questa legislatura che torniamo e lo attraversiamo perché è un tema importante che lo si ritrova in tutta la Costituzione. Nell'articolo 13 viene sancito con estrema chiarezza, però vorrei sottolineare quando lei ha parlato di responsabilità del contesto. La politica non può essere lo spazio per comodi accessi al consenso e questa è la responsabilità del contesto, sempre. Noi anche durante la pandemia abbiamo occupato questo spazio scomodo della politica. Non è stato semplice e oggi i fatti ci dimostrano che, purtroppo, avevamo ragione. Allora, noi siamo contro l'affermazione che bisogna marcire in galera. In galera non si marcisce; se si ha l'idea che chi va in galera marcisce, questo è l'impianto da rovesciare e cambiare. È questo il senso dell'articolo 27 della Costituzione, dell'articolo 13 e di tutta la Costituzione, ma è questo il senso della sicurezza, cui tutti noi teniamo. La sicurezza è legalità fuori dalle carceri come dentro le carceri. La sicurezza è un concetto di protezione e di tutela. È ancora più grave quando chi è il tutore della libertà e della nostra sicurezza si macchia di questi fatti molto gravi essendo in una posizione di autorità. Non possiamo accontentarci, pertanto, di parole postume di vicinanza o di impegni astratti e la ringrazierò per le sue parole e per averci richiamato alla responsabilità del contesto. Ci sono molte cose da fare. C'è da riprendere la riforma dell'ordinamento penitenziario, investire sul trattamento, sul personale e sulle risorse perché le carceri siano più umane anche per chi ci lavora. Se non vogliamo retoricamente rivolgerci indossando qualche felpa o qualche mezza divisa a seconda delle stagioni e se vogliamo parlare sul serio anche ai custodi penitenziari, dobbiamo occuparci delle condizioni delle carceri delle carceri e del fatto che la pena sia modulata a seconda del percorso e che non ci siano automatismi. Anche questo non è da oggi che lo scopriamo. Ci siamo battuti per eliminare tutti gli automatismi sulla pena e sugli aggravamenti di pena e continueremo a batterci perché questa è la strada da battere. Allora, diciamo sì a più risorse, più spazi per il trattamento, la rieducazione e per la formazione anche degli agenti penitenziari, sempre per sfuggire dalla comoda retorica dell'attenzione a questo o a quello. Sugli sconti di pena, è già così: chiunque frequenti un carcere o un tribunale di sorveglianza sa che c'è un'osservazione del detenuto, ma il punto è che ci sono pochi psicologi, pochi assistenti, c'è poco personale dedicato a questo. Abbiamo

non a correnti alternate. Il garantismo è un concetto globale, è la legalità nel processo, è la legalità nelle sanzioni, è la legalità nelle carceri. Ridiscutiamo

perché le sue parole sono state parole di verità e senza reticenza. Per questo la ringrazio davvero, perché abbiamo segnato in questo momento, in quest'Aula, grazie a lei, un primo passo e ha fatto bene a ricordare questa coincidenza con il 21 luglio di vent'anni fa. Accadde ieri, è accaduto oggi, non deve più accadere. Abbiamo ascoltato con attenzione la sua informativa sull'orribile mattanza avvenuta il 6 aprile di un anno fa nel reparto Nilo, dove 292 detenuti sono stati vittime di violenze, di una pluralità di azioni contrarie alla dignità e al pudore, degradanti e inumane, inaccettabili per uno Stato di diritto. Quando lei è andata a Santa Maria Capua Vetere si è accorta che mancava l'acqua corrente. Lo Stato deve fare autocritica: lo sa che quel carcere è stato costruito con le aziende della camorra casalese? Così è stata messa in piedi una struttura dello Stato e non sono i retroscena giornalistici, ma ci sono inchieste della magistratura. Siamo tutti preoccupati, altro che perquisizione straordinaria e generalizzata, è stata davvero una mattanza organizzata nei minimi dettagli e con la copertura evidentemente della catena di comando. Se lei ha ricordato il 21 luglio di vent'anni fa una ragione ci deve essere stata. Per questo, con altri colleghi, con la senatrice Valeria Fedeli e con il senatore Franco Mirabelli chiediamo al Senato, al Presidente e ai Gruppi, di una Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema del carcere a 360 gradi, perché non c'è ombra di dubbio che i detenuti siano vittime di violenze, ma non c'è ombra di dubbio che anche il personale penitenziari viva in condizioni drammatiche. Ci sono realtà in cui è applicata la funzione rieducativa della pena ed è osservato il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, ma c'è bisogno di risposte immediate alle tante domande che ognuno di noi si pone dopo aver visto quelle immagini scioccanti, che hanno spinto proprio lei ad affermare che è stata tradita la Costituzione. Le scene diffuse nei giorni scorsi si riferivano a quindici mesi fa; nel frattempo in quel penitenziario hanno vissuto insieme gli stessi agenti e gli stessi detenuti, anche se l'allarme era stato lanciato nell'immediatezza, poi abbiamo sentito dell'interrogazione parlamentare. È questo il *vulnus.* Perché il Ministero, il DAP, non è intervenuto? Certo, poi le immagini sono state sequestrate dalle inchieste della magistratura, c'è il segreto istruttorio, per cui ne siamo venuti a conoscenza un anno dopo perché la magistratura ha i suoi provvedimenti restrittivi.

uccisi per difendere la legalità. *(Applausi)*. Mi piace ricordare il vice direttore del carcere di Poggioreale Giuseppe Salvia, l'agente Pasquale Campanello, l'educatore del carcere di Opera Umberto Mormile. Lei ha parlato di un detenuto con la tua fragilità, la salute mentale, i problemi. Ci sono le questioni sanitarie. Abbiamo bisogno di più agenti perché sono soli, pochi e malpagati. Abbiamo bisogno di formazione, di più educatori, di più assistenti sociali. Mai più fatti come quelli avvenuti. Signor Presidente, Ministro, colleghi, mi unisco certamente ai ringraziamenti al Ministro sia perché ha avuto la sensibilità di venire alle Camere sia soprattutto per quello che ha detto. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi. Vorrei pormi una domanda, che rivolgo collettivamente, ovvero che cosa può fare oggi concretamente il Parlamento per dare delle risposte. Mi sono data anche una risposta perché nelle stesse parole del Ministro c'è una risposta, se volete, pragmatica e concreta. Gli interventi che si possono fare in termini di edilizia giudiziaria sono collegati al *recovery*, quindi, questo Parlamento, se vuole concretamente fare qualcosa perché si migliorino le nostre carceri, gli edifici, le condizioni di vita, deve assumersi la responsabilità di fare quello che peraltro si è già impegnato a fare, e cioè approvare rapidamente le riforme chieste dall'Unione europea in materia di giustizia.

ma abbiamo il dovere di rispondere con atti concreti, ovvero dare seguito all'impegno che il Governo, e in prima persona il Presidente del Consiglio ha assunto in ordine alle tempistiche di approvazione delle riforme. Questa è la nostra responsabilità collettiva, e questo è quello che dobbiamo fare prima di tutto. Anche perché l'edilizia giudiziaria

Mi permetto anche di dare un piccolo contributo, volendo ricordare che gli attori all'interno del carcere sono tanti. Giustamente si è detto che non si deve colpevolizzare la polizia penitenziaria perché fa un lavoro terribile in condizioni terribili, ma non dobbiamo neanche dimenticare l'opera che svolgono i funzionari giuridici pedagogici e gli assistenti sociali, che sono il tramite tra i detenuti e la magistratura, soprattutto quella deputata. Dobbiamo anche ricordare che una riflessione collettiva sull'esecuzione della pena è stata fatta con gli stati generali dell'esecuzione penale. Lo ha ricordato giustamente il Presidente delle camere penali. È stata una riflessione che ha dato una serie di indicazioni su un tema sicuramente scottante e complesso, che andrebbe ripreso, perché i fari richiamati dal Ministro e dai tanti interventi, che dobbiamo sempre tenere presenti, sono, da una parte, le norme costituzionali, ma, dall'altra - permettetemi - il monito

degli agenti penitenziari e allora è oscillato tutto da un'altra parte; poi si è parlato del fatto che dal carcere uscivano i mafiosi e si è oscillato di qua,

fare un *focus*, che beneficia anche della sensibilità da sempre dimostrata dal Ministro su questi temi. Santa Maria Capua Vetere rappresenta la cifra estrema di quello che abbiamo visto tragicamente, di tutto quello che è stato rappresentato.

si parla di Costituzione tradita, di responsabilità collettiva, di un sistema che va riformato. Ci attendiamo però che a questo punto, e da questo momento in avanti, anche in vista della della prospettiva europea, che alle parole seguano i fatti, perché il carcere e l'esecuzione penale nel suo complesso siano plasmati in una maniera efficace e definitiva verso un sistema rispettoso della dignità, dei diritti fondamentali e realmente teso alla risocializzazione del reo. Oltre a quanto immaginato dal Governo, con il Piano nazionale di ripresa e con l'impiego delle risorse straordinarie europee sul versante strutturale del carcere, è giunto il momento di una riforma complessiva. Non si tratta soltanto di implementare nuove carceri, ma occorre con forza realizzare un carcere nuovo, cioè rinnovato quanto ad assistenza, trattamento, produttività e formazione per renderlo finalmente conforme alla nostra Carta costituzionale.

una frase chiara, che non si presta a pluralità di interpretazioni. Il sistema penitenziario è riuscito solo in poche occasioni a rispettare tali imperativi costituzionali e normativi e, nonostante i tanti anni trascorsi, i luoghi di detenzione hanno costituito sempre sempre una spina nel fianco nel nostro Stato di diritto, che nessuno è riuscito a estirpare, nonostante la sottoscrizione di Trattati internazionali, raccomandazioni e condanne diverse provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiaramente alcune linee di intervento sono emerse. Il Ministro ha parlato in maniera molto chiara di interventi sulle strutture, sul personale e sulla formazione. Penso anche al nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario dell'ordinamento penitenziario del 2000, che andrebbe riscritto, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel mondo esterno, della riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore nell'ottobre del 2018, degli insegnamenti appresi dalla crisi sanitaria e della necessità di rendere il carcere un luogo responsabilizzante, nel quale la vita scorra nel modo più simile possibile a quella esterna, in vista di un ritorno in società delle persone detenute. Più risorse anche per le misure alternative per la giustizia di comunità, progetti educativi e sociali che riducano i rischi della devianza, trattamenti socio-terapeutici esterni per chi ha problemi di dipendenza. Più risorse per modernizzare e migliorare la vita interna. Le ristrutturazioni sono necessità non più rinviabili, così come il potenziamento di strutture mediche ed infermieristiche. Più risorse da investire nel capitale umano; gli educatori presenti sono il 18 per cento in meno di quelli previsti: 733 invece di 896. Questo vuol dire un educatore ogni 73 detenuti. Il trattamento economico a loro riservato è nettamente inferiore rispetto a quello degli agenti. I funzionari amministrativi sono il 21,6 per cento in meno di quelli previsti. Ugualmente medici, infermieri, psicologi sono insufficienti, al pari degli assistenti sociali. Con il *recovery* arriveranno in Italia oltre 200 miliardi di euro. Una parte andrà alla giustizia e al sistema penitenziario. È davvero un'occasione da non sprecare con una serie di interventi che analiticamente sono stati già delineati in sede di rappresentazione delle linee guida e delle linee programmatiche del Ministro in Commissione giustizia; siamo certi che vi daremo seguito in questa fase così delicata e in uno snodo essenziale per la vita del Paese.

con 160 articoli circa. Un decreto-legge che utilizza una cifra di circa 40 miliardi, che poi è l'importo dell'ultimo scostamento, ultimo di una serie di scostamenti che hanno incrementato

una specie di mostro, come ormai siamo abituati a vedere, valutare e considerare: una specie di mostro normativo che spazia. Una volta c'erano i mille proroghe; poi gli *omnibus*, poi

un decreto-legge che proroga e ripropone pezzi di decreti emergenziali della coppia Conte-Arcuri, tanto per confermare che, in gran parte dei suoi provvedimenti concreti, questo Governo altro non fa che rimettere mano, quasi sempre senza determinare grandi mutazioni, a provvedimenti già adottati dal precedente Governo Conte. Gli esempi non mancano. Gli esempi non mancano. Colleghi, come sapete, io cerco di occuparmi soprattutto di temi sanitari. In questo decreto ci sono molti articoli che trattano della materia, in questo momento, peraltro, particolarmente sensibile rispetto alla vita quotidiana degli italiani. Ebbene, il comma 2 dell'articolo 26 rimette mano

in tempi di Covid-19. Si tratta di circa 50 milioni, più o meno, di prestazioni, tra diagnostica e trattamenti sanitari rimasti in sospeso, che le Regioni devono recuperare. Sono state destinate risorse, con due successivi provvedimenti legislativi, praticamente in fotocopia,

viene solo prorogato il termine per rendicontare, ma non cambiano i criteri per l'utilizzo di queste risorse e soprattutto per il piano di riparto delle risorse tra le Regioni, che non tiene in alcun conto

500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. qui già serve il traduttore. Poi però si spiega che, per i profili inerenti al settore sanitario,

anche privati per il sequenziamento di nuova generazione, definito con un acronimo. Abbiamo un problema serio

prevedere un provvedimento legislativo che aumenti la nostra capacità di sequenziare, ma il problema, colleghi, è che non serve chissà cosa per sequenziare. Bisogna però spendere denaro e comprare i sequenziatori, che esistono sul mercato e vengono forniti da numerosi operatori. Se riteniamo che, per un provvedimento che intende incrementare la nostra capacità di sequenziare, è sufficiente investire 46 milioni di euro per il 2021 e 23 milioni di euro per il 2022 significa che siamo veramente molto ottimisti, al limite dal poter

C'è invece una cifra corposa, che non è per nulla chiarita, a disposizione del commissario straordinario, pari a 1.650 milioni di euro, per il 2021 e quindi - attenzione! - per uno scorcio di anno.

Temo che questa cosa rimanga nell'immaginazione collettiva; noi non sappiamo che cosa accade in questo momento. Ci mancherebbe, nessuno di noi se la sente di criticare l'operato del generale, ma vorremmo capire perché abbiamo abbattuto così drasticamente la quantità di vaccini somministrati. E non è pensando di introdurre un obbligo surrettizio al vaccino, quale quello del *green pass*, che possiamo pensare di risolvere questo enorme problema. Questo enorme problema lo dobbiamo affrontare con una campagna seria di informazione e coinvolgendo adeguatamente i medici di medicina generale; insomma, con provvedimenti di sistema

di una critica spinta nei confronti dell'ennesimo provvedimento che viene portato a scatola chiusa, senza la possibilità di modificare nulla e senza la possibilità di migliorare neanche le cose più

Si tratta di un provvedimento imponente, nato con l'intento prioritario di puntellare il tessuto economico e sociale del nostro Paese, fortemente fiaccato da questo ormai anno e mezzo di pandemia. Attenzione: se questo Governo, in questa fase, riesce a finalizzare misure di tale portata, è anche grazie al grande lavoro che è stato fatto a partire dal febbraio 2020. Quello del decreto sostegni-*bis* è solo un capitolo della saga, dal cura Italia al decreto liquidità, dal decreto rilancio al decreto agosto, passando per tutti i vari decreti ristori. Il solco su cui poggia il puntellamento del nostro sistema economico è stato tracciato da un signore di nome Giuseppe Conte a cui deve andare il nostro più sentito ringraziamento per come ha saputo imbastire questo immane lavoro nell'ora più buia per il nostro amato Paese. Quindi chiariamo subito che, se oggi riusciamo a ottenere molto per le nostre imprese, per le nostre famiglie per il nostro sistema sanitario, è anche grazie a quanto di buono è stato seminato durante il 2020. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il decreto-legge sostegni-*bis* punta a dare una spinta alle attività produttive del nostro Paese. Sono quasi 15 e mezzo i miliardi destinati a fondo perduto alle piccole e medie imprese, ai commercianti, agli artigiani, agli operatori turistici, agli agricoltori e a tantissimi altri comparti produttivi. La novità principale è che, di questi 15,4 miliardi, oltre 3 sono dedicati alle imprese che decidono di calcolare la loro perdita di fatturato dall'aprile 2020 invece che da gennaio. Altri 4 miliardi invece verranno erogati sulla base del risultato di esercizio, tenendo conto dunque dei bilanci consuntivi e non del fatturato. Dopo aver superato i codici Ateco, strumento che purtroppo si è reso necessario, ma che non ha contribuito a semplificare la vita degli italiani, abbiamo raddrizzato lo scenario anche sul fronte del fatturato, grazie al grande lavoro fatto dal MoVimento 5 Stelle durante l'*iter* parlamentare del provvedimento. Poi siamo riusciti a prorogare per altri cinque mesi il credito di imposta per gli affitti a uso commerciale per quelle attività che hanno visto andare in fumo oltre il 30 per cento del proprio fatturato. Abbiamo prolungato ulteriormente anche lo sconto sulle bollette energetiche per le nostre imprese e finanziato con 600 milioni di euro per l'anno 2021 una riduzione della Tari da parte dei Comuni in favore delle categorie colpite dalle chiusure. Per il settore sportivo è prevista la riproposizione per tutto il 2021 del credito d'imposta al 50 per cento sugli investimenti pubblicitari delle realtà sportive che investono nei settori giovanili, così come già precedentemente previsto per quelli effettuati nel secondo semestre del 2020. In più, si è incrementato con ulteriori 180 milioni di euro per tutto il 2021 il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. in esame mettiamo un argine anche all'emorragia di giro d'affari di settori cruciali come quelli del tessile, della moda e del *wedding.* È prevista la proroga per tutto il 2021 del credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino per le imprese del tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

previsto un altro fondo da 50 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare contributi in favore di iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici dei Comuni in cui sono ubicati i siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Abbiamo voluto prolungare anche il credito d'imposta del 65 per cento per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. signor Presidente, mi faccia esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto sul fronte delle compensazioni per quelle imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche che si trovano a dover combattere con oscillazioni folli dei prezzi dei materiali. La pandemia, tra le tante sciagure, ci ha portato in dote anche rincari indiscriminati di tantissime materie prime e, per questo aspetto, si sta rivelando una vera e propria zavorra per moltissimi segmenti produttivi. Dopo aver fatto questo sforzo immane per dare precise garanzie a chi opera nel settore delle grandi infrastrutture, è necessario individuare il prima possibile strumenti per aiutare altri settori, anche all'interno dell'edilizia stessa. quando il sottosegretario Fraccaro iniziò a ipotizzare l'idea di un superbonus al 110 per cento per la riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico degli edifici privati, alcuni in quest'emiciclo ci presero per pazzi visionari. Ora, invece, tutte le forze politiche sono ben consapevoli di quanto quel meccanismo fiscale sia una locomotiva cruciale per la ripartenza della nostra economia e, in particolare, del settore dell'edilizia. una misura che dà concretezza a un termine - quello della transizione ecologica - sul quale per ora questa maggioranza ha saputo produrre soltanto tante chiacchiere e pochissimi contenuti. contenuti. Mi preme sottolineare, però, un comportamento davvero disdicevole, che non può essere sottaciuto in alcun modo: mentre nelle Commissioni e nelle Assemblee parlamentari ci sforziamo di dare il massimo per formulare e migliorare decreti colossali come quello oggi al voto, fuori c'è gente che si attiva per abolire il reddito di cittadinanza e non per reale convinzione politica. I signori che blaterano certe fesserie, cannoneggiando il reddito di cittadinanza, lo fanno non certo per ideologia o perché hanno un'alternativa, ma solo per andare contro il MoVimento 5 Stelle e per interessi piccoli di consenso e bottega. A questi signori non importa nulla se i percettori del reddito di cittadinanza, nei mesi più difficili della storia repubblicana, sono riusciti a mettere in fila il pranzo con la cena. A questi signori non importa nulla se il nostro Paese ha uno dei tassi di povertà più alti dell'Unione europea,

Diciamo una volta per tutte che il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo, ma dignità: quella dignità che chi chiede di abolirlo dimostra di non avere. Non dedico che poche righe a chi obietta che vi sono dei percettori abusivi che non ne hanno diritto. Bene, quando scoperti, la legge farà il suo corso. Pensate che tutte le pensioni di invalidità siano dovute o che qualcuno sotto Naspi non sia scorretto? Vanno incentivati i controlli e puniti i comportamenti illegali, ma non per questo si può mettere in discussione questo provvedimento. Lo ha pensato il MoVimento 5 Stelle e per questo deve essere demolito. Ma basta, basta. La Meloni, senza vergogna, lo definisce metadone per tossici. Ma si possono sentire dichiarazioni di questo tenore? No, non si possono sentire. Ringraziate che la vita non vi abbia posto in situazioni di difficoltà. mio intervento dicendo: portiamo a casa questo decreto-legge che tocca milioni di italiani in diversi modo (insegnanti, medici, infermieri, negozianti, piccoli e grandi imprenditori, ristoratori, proprietari di palestra e tanti altri ancora). Smettiamola una volta per tutte di prendercela con chi non ha nulla e la notte perde il sonno pensando a come arrivare a fine mese. Sarebbe un atto di maturità per tutti e qui l'età della maturità ce l'abbiamo davvero tutti.

ancora più svantaggiate. Vi dovrei fare l'elenco di tutti i provvedimenti che sono stati valutati, ma mi riservo di dire che si tratta delle categorie veramente più svantaggiate: parlo ad esempio delle partite IVA. Chi di voi non conosce una persona con una partita IVA che in questo periodo purtroppo ha avuto dei grossi problemi? Mi riferisco anche - l'ha anticipato il collega Lanzi, ma mi aggiungo - al reddito di emergenza: con tutte le critiche, abbiamo comunque salvato delle persone e delle famiglie che hanno sofferto tantissimo

ordini del giorno con i quali abbiamo posto l'attenzione davvero sul bisogno psicologico delle persone. È su questo che vorrei soffermarmi in particolar modo, sulla battaglia che abbiamo fatto come PD, con la nostra capogruppo Simona Malpezzi, che ha voluto un ordine del giorno che si è tramutato in un emendamento importante alla Camera. Abbiamo messo a disposizione dei fondi per finanziare il sostegno psicologico per i figli, gli adolescenti e le famiglie, che hanno bisogno di essere supportati in questo periodo terribile. Sono stati messi a disposizione dei fondi per assumere psicologi nel sistema sanitario nazionale, per assicurare prestazioni psicologiche, anche domiciliari,

La resilienza di cui tanto ci riempiamo la bocca si costruisce insieme ai professionisti che ci guidano per poterlo fare. Quindi, questi diritti devono essere garantiti. Un altro

pre-Covid, avevamo grossi problemi, però è importante che siano state fatte piccole azioni di concretezza. Non meno importante è il supporto alle persone più fragili, come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche: anche su questo abbiamo fatto una grande battaglia, anche con mozioni, andando a rivedere quel nuovo piano oncologico, in cui davvero

i colleghi lo sanno molto bene - a quello che dovremo affrontare con le perdite di lavoro che ci saranno prossimamente: mi auguro che il Governo saprà affrontare tutto questo. Finora lo abbiamo fatto con la programmazione dei licenziamenti più avanti e con le proroghe,

emendamento, che mi ha vista partecipe con la prima firma già nei precedenti provvedimenti, non era mai riuscito purtroppo, per motivi di inammissibilità, ad arrivare a buon fine. Alla Camera ci sono riusciti e ora mi auguro che sia definitivo. Abbiamo recepito l'appello di tantissimi operatori sociosanitari, affinché questo emendamento arrivasse alla fine del suo processo. Oggi possiamo dire che siamo certi che questa cosa è avvenuta e ce ne facciamo carico.

ma se non rafforziamo il nostro personale, i professionisti, se non diamo loro le competenze e non diamo loro anche le motivazioni per andare avanti, come il riconoscimento di questo ruolo, credo che non faremo un grande lavoro. Io penso che la sanità abbia bisogno di strumenti, di tecnologia e soprattutto del fattore

decreto-legge sostegni-*bis* soprattutto per la parte che riguarda l'istruzione perché mi pare che sul resto sia stato detto molto. Certo, ci sono diverse criticità che riguardano lo sblocco dei licenziamenti, per esempio, che purtroppo sta mettendo in grave crisi migliaia di lavoratori. È una cosa estremamente grave,

anche a tutti coloro che avrebbero dovuto affrontare il concorso ordinario. Sono tre anni ormai che gli aspiranti docenti aspettano il concorso ordinario. È dal 2018 che ci stiamo lavorando, ma le forze politiche sul concorso ordinario, le cui procedure selettive possono riguardare tutti e sono previste dalla Costituzione,

ma per i requisiti di accesso si creano corsie preferenziali, creando dei percorsi non selettivi di reclutamento per alcuni,

Tutte le procedure ordinarie sono sospese *sine die*; non si sa quando verranno riprese, mentre vengono varate quelle straordinarie, che si sovrappongono ad altre che si sono appena concluse. Quindi, ancora più posti andranno ai cosiddetti precari, tra cui molti, purtroppo, non sono neanche abilitati. Anche per loro è stata attivata un'ulteriore procedura differenziata dalle altre. Mi domando: se tutti dovranno essere docenti, tutti si dovranno sedere in cattedra, tutti avranno lo stesso stipendio, per quale motivo si creano percorsi differenziati quando i requisiti per insegnare devono essere gli stessi? Perché si vuole continuamente non solo insidiare il dettato costituzionale, ma anche creare delle situazioni in ingresso che pregiudicano anche la qualità della formazione dei nostri studenti, che è l'aspetto al quale dovremmo guardare prioritariamente. Invece, purtroppo, non lo facciamo perché su quello non c'è alcun impegno, se non solamente nominale. Basta pensare al piano estate, che si basa soltanto su attività ludico-ricreative e di supporto e sostegno psicologico, mentre nulla si fa

a creare e a formare cittadini liberi, consapevoli e dotati di coscienza critica. Purtroppo i dati Invalsi ci restituiscono, invece, un quadro totalmente diverso e se a fronte di ciò non ci porremo le domande necessarie per un ripensamento del nostro sistema di istruzione in una direzione ben

presi dalle graduatorie per le supplenze, che non sono fatte per dei percorsi di reclutamento. Nel momento in cui i docenti verranno avviati nei percorsi di reclutamento, poi dovranno rimanere nelle Regioni dove hanno fatto richiesta per tre anni, perché si vedranno applicato il blocco della mobilità. Anche questa è è una cosa che non condividiamo affatto. Ci sono stati dei miglioramenti rispetto al testo che era stato varato dal Consiglio dei ministri, ad esempio abbiamo visto che è stato ripristinato il regolamento per il concorso per dirigenti tecnici, ma ci auguriamo anche che venga bandito immediatamente, ci sono soltanto 35 ispettori scolastici e dirigenti tecnici in tutta Italia e non si può continuare così, perché le scuole sono in balia di sé stesse e di abusi di tutti i tipi,

grazie al quale quantomeno per l'accesso a questi finanziamenti le scuole dovranno rendere pubblici i bilanci e gli organici, cosa che speriamo eviterà che le risorse vadano anche ai tanti diplomifici che ci sono in tutta Italia. Ma questo dovrebbe valere anche per la parità scolastica, che dovrebbe essere concessa solo a determinate condizioni, cioè a condizione che questi istituti abbiano bilanci pubblici e trasparenti e organici pubblici e trasparenti: solo così si può accettare che delle scuole private possano essere equiparate a quelle dello Stato, così come i titoli di studio. Ci sono ancora

nell'affrontare le risposte all'emergenza e per la ripresa del Paese, questo Governo ha evidentemente segnato un coraggioso cambio di passo rispetto al precedente.

senza un ordine di reale priorità, svilendo l'efficacia delle tante risorse comunque messe a disposizione, troppo spesso sprecate dal Governo Conte. primo decreto sostegni ha fatto seguito il decreto sostegni-*bis*, la cui organicità al primo è data dalle misure inserite nel decreto, anche dando seguito agli ordini del giorno che proprio in quest'Aula erano stati votati come impegno preciso al Governo per il sostegni-*bis*. Come relatrice di maggioranza al primo decreto sostegni, esprimo soddisfazione perché il lavoro del Senato non si è esaurito con il primo provvedimento, ma è continuato anche in questo decreto-legge. Nonostante la seconda lettura in Senato abbia trovato tempi molto compressi e l'impossibilità di qualsiasi modifica, questo ramo del Parlamento si è comunque potuto esprimere attraverso ordini del giorno impegnativi, ed è stato preso in considerazione dall'Esecutivo. Ogni ordine del giorno si è trasformato in norma, e lo stesso auspichiamo possa avvenire per quelli odierni. Fondamentali, pertanto, sono le risposte date per la copertura dei costi fissi su cui ci eravamo molto impegnati, per le attività che hanno subito chiusure, che vanno a completare le misure adottate nel decreto-legge sostegni, come il credito d'imposta per i canoni di locazione, l'esenzione della Tari, ulteriori fondi per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e fondi a sostegno delle attività e dei settori maggiormente penalizzati dalla crisi. contempo, ci eravamo impegnati per ulteriori indennità per i lavoratori stagionali e dello sport, per la moratoria sui prestiti fino al 31 dicembre 2021, per la proroga e la rimodulazione degli strumenti di garanzia. Sia attraverso i contributi a fondo perduto sia attraverso l'accesso al credito, non si deve lasciare indietro nessuno, pena la messa in discussione di un sistema di indotto su cui poggia in modo particolare il nostro Paese. Ad esempio, pensiamo a un settore fortemente penalizzato dalla crisi e che rappresenta un importante componente del nostro PIL, ovvero il turismo. Non dobbiamo dimenticare che questo costituisce in maniera diretta il 6 per ma arriva al 13 per cento, quindi più del doppio, grazie a tutto l'indotto a esso collegato. Togliere un tassello del nostro tessuto produttivo rischia di far crollare gran parte del sistema. In questo momento storico gli equilibri sono molto precari. Alla crisi dettata dalla pandemia e alle conseguenti chiusure si aggiunge ora la mancanza delle materie prime e l'aumento incontrollato dei costi delle stesse, che stanno creando maggiori difficoltà alle imprese, ma anche ai sindaci. Pensiamo alle opere pubbliche, in particolare penso all'edilizia scolastica: è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno *ad hoc*. Pensiamo al settore dell'*automotive*: sta impattando ora sui ricavi e sui volumi l'interruzione della produzione proprio a causa della mancanza di chip e di materie prime. Questo, tra l'altro, è uno di quei settori a cui la Commissione europea chiede una riconversione per eliminare le emissioni di CO2 entro il 2035. Quindi, bene lo stanziamento di 350 milioni a sostegno del settore, con 15 milioni di risorse dedicate all'acquisto dei veicoli elettrici, quindi un prolungamento dell'ecobonus. Siamo in una fase cruciale, andare oltre le misure emergenziali, per garantire stabilità a tutti i settori in previsione anche della transizione. Una transizione che deve avere tempi adeguati e garantire contemporaneamente sostenibilità economica e sociale, e questo Governo ha dato prova di saper rispondere, senza rincorrere solo il virus, alle esigenze del Paese. *(Applausi)*. che Forza Italia sostiene la necessità di una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro; finalmente, con il decreto sostegni-*bis* si è messo in discussione in maniera strutturale il decreto-legge dignità, aprendo ai contratti a tempo determinato, almeno fino alla conclusione del 2022, benché attraverso la contrattazione collettiva. Servono, infatti, maggiori opportunità, che sono date anche attraverso la flessibilità e soprattutto potenziando e riorganizzando la formazione. Il processo di cambiamento lo richiede, e in questo senso il Piano nazionale di ripresa L'occupazione va garantita attraverso la formazione, il sostegno al sistema impresa, gli investimenti, regole certe, le riforme. Il blocco dei licenziamenti è stato utile per garantire la coesione del sistema sociale nei momenti più cruciali di questa pandemia. Tenere, però, la linea esclusivamente in questa direzione non avrebbe che incancrenito il problema. Le aziende che irresponsabilmente hanno licenziato circa 570 lavoratori senza se e senza ma, senza nemmeno consentire di usufruire degli ammortizzatori sociali e di concordare un tavolo con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, non incarnano i valori etici e morali della stragrande maggioranza dei nostri imprenditori. Bisogna intervenire, non c'è più tempo da perdere, per evitare le delocalizzazioni di massa che, ricordo, avrebbero dovuto essere fermate sempre con il cosiddetto decreto dignità. Tra gli obiettivi originari del decreto citato uno era quello di abolire il precariato, l'altro di penalizzare le aziende che avessero delocalizzato. Ricordo che, pur a fronte di un aumento dei contratti a tempo indeterminato nel 2019 rispetto al 2018, l'Osservatorio sul precariato dell'INPS ha rilevato una diminuzione dei posti di lavoro: 876.000 nel 2018, 842.000 nel 2019. quindi evidente che pur a fronte di una diminuzione del precariato, è aumentata la disoccupazione. Non è trattenendo le imprese all'interno dei confini nazionali con gravosi meccanismi sanzionatori che si mantengono i posti di lavoro o se ne producono di nuovi. L'abbiamo purtroppo visto e l'avevamo previsto. I tavoli di crisi sono fermi al 2018. Troppo e male ci si è impegnati per il reddito di cittadinanza e troppo poco per le imprese. affermava che «se l'impresa è sveglia, la ricchezza si accumula, non importa quel che faccia il risparmio; se l'impresa dorme, la ricchezza decade, qual che sia la sorte del risparmio». Ora si apre uno scenario in cui si deve avere il coraggio di cambiare, di modificare quello che non va bene, di abbandonare le proprie di ideologie e di remare tutti insieme verso il 2026, il 2027, il 2035 e il 2050. La transizione energetica avrà sicuramente bisogno di più tempo per concludere il processo rispetto a quanto previsto dall'Unione europea. Queste date segnano però obiettivi di grande respiro per il nostro Paese per stare al passo e non solo perché lo richiede l'Europa, ma perché ce lo chiede il nostro sistema Paese.

noi di Fratelli d'Italia questo metodo non potrà mai andar bene; fatevene una ragione. Ormai non siamo più in un bicameralismo perfetto, lo chiamerei un monocameralismo a fasi alterne; una volta fate discutere i provvedimenti alla Camera, un'altra volta li fate discutere al Senato. Insomma, anche nelle Istituzioni si fanno i turni, a causa purtroppo del protagonismo del Governo,

Il problema è che voi mettete la fiducia perché avete una maggioranza unita solo da due questioni: la voglia di poltrone e di potere,

il provvedimento è come una manovra finanziaria colleghi perché ha un valore di 40 miliardi di soldi degli italiani e quindi per noi è assolutamente ingiusto che non ci sia un dibattito. Si tratta infatti di debiti che peseranno e graveranno sui nostri figli. Ormai questo atteggiamento continua a ripetersi da molto tempo. Io però lo faccio un appello alla presidente del Senato; credo infatti che la presidente del Senato dovrebbe attivarsi perché sia ripristinata la piena agibilità democratica. Non mi sembra che siamo in queste condizioni.

D'altra parte, cosa ci possiamo aspettare da una maggioranza che litiga assolutamente su tutto, da una maggioranza che in queste ore parla di *green pass* obbligatorio per andare allo stadio e forse anche per prendere il caffè? Vorrei però sapere Vorrei però sapere se anche gli immigrati che arrivano irregolarmente sulle nostre coste dovranno essere dotati di *green pass* o se il vostro accanimento terapeutico è solo ed esclusivamente sugli italiani, sui lavoratori, sugli imprenditori, sulle aziende.

e sarà commisurato al vostro fallimento nella gestione disastrosa sia di questa pandemia nella vita quotidiana, sia del nostro sistema economico. Capisco che anche adesso voi cerchiate forse di rendere obbligatorio il vaccino, perché voi siete così:

A mio avviso questo Governo e questa maggioranza vivono alla giornata perché non hanno un orizzonte futuro, lo dico a ragion veduta. Voi pensate veramente che tutti i problemi della nostra Nazione si possano risolvere attraverso la decretazione d'urgenza? No, signori, non è questo il modo. Credo che ci sia un'urgenza nel nostro Paese ed è quella di mandarvi a casa il più presto possibile, perché fate tante chiacchiere, pochi fatti e siete anche degli ipocriti. Vi dite preoccupati per la fine del blocco dei licenziamenti, però poi bocciate le proposte di Fratelli d'Italia per dimezzare il costo del lavoro. lavoro. Abbiamo visto in questi giorni che vi ergete a paladini dei diritti LGBT e poi siglate accordi commerciali in quei Paesi dove l'omosessualità è un reato punito addirittura anche con la pena di morte. Lasciate che gli italiani si assembrino ovunque, nelle strade, nei *gay pride,* nei *rave party*, ma vi ostinate ancora a tenere chiuse le discoteche. Ripetete di essere aperti al confronto con le opposizioni: chi di voi va in televisione dice che voi siete per il dialogo, siete aperti con le opposizioni, ma poi in realtà bocciate in maniera sistematica tutte le tutte le proposte di buon senso avanzate da Fratelli d'Italia. Vi definite democratici, ma poi bloccate il Parlamento, imbrigliando il dibattito, e l'unica cosa che vi viene benissimo - mi rivolgo al Governo

ieri abbiamo discusso ampiamente del disegno di legge Zan. Peraltro, l'ampia discussione non è ancora conclusa. Ieri, nel mio intervento, vi ho parlato di priorità priorità per il nostro Paese. Il provvedimento che andiamo a discutere oggi, molto velocemente, peraltro, e con tempi ridotti dall'imminente scadenza, rappresenta, nella mia scala di priorità, una priorità. In Senato ci eravamo occupati del primo decreto sostegni, con cui avevamo dato inizio a una nuova stagione di aiuti alle imprese, alle famiglie, alle partite IVA e alla ripresa dell'economia dopo le chiusure forzate dovute alla crisi sanitaria.

tanto è vero che molte erano rimaste le questioni irrisolte, messe in evidenza da un ordine del giorno, concordato tra noi senatori e firmato dai Capigruppo di maggioranza. Quell'ordine del giorno,

Quindi, colleghi, possiamo comunque ritenerci soddisfatti per aver svolto un buon lavoro preparatorio. Oggi, però, ci troviamo ad esaminare velocemente questo testo, lavorato ed implementato dai colleghi della Camera. Camera. Quando si tratta di lavorare sodo su questioni concrete, la Lega dimostra sempre il pragmatismo delle sue donne e dei suoi uomini. Ed è per questo seppur per noi al Senato il tempo di analisi sia stato molto ristretto, voglio ringraziare i componenti del Gruppo Lega della Commissione bilancio per il grande lavoro svolto alla Camera e per i risultati ottenuti. In particolare mi congratulo con il relatore, Massimo Bitonci, che ha reso possibile l'inserimento, nell'articolato originario, di parecchi emendamenti fortemente voluti dalla Lega e concordati con tutta la maggioranza. L'elenco è già stato abbondantemente citato dalla collega Faggi, ma è giusto anche ricordare tutti gli interventi su tasse, proroghe, fiere, terzo settore, settore Horeca e *wedding*; e poi interventi su imprese, con rifinanziamento della legge Sabatini, sul settore terme, sul settore agricolo, con il fondo gelate, sul settore apistico e sull'*automotive*, con l'estensione degli incentivi anche per l'acquisto di veicoli usati con basse emissioni. Questa è una novità. Ancora, interventi per le guide turistiche e per i bus turistici, interventi sullo sport, con contributi a fondo perduto anche su impianti sportivi, in particolare sulle piscine, altri interventi che non sto qui ad elencare. Questi, forse, sono gli interventi che più mi stanno a cuore. Un passo avanti è stato fatto anche verso i proprietari di immobili colpiti dal blocco degli sfratti, con l'estensione a tutto il 2021 dell'esenzione dal pagamento dell'IMU. Allo stesso modo è stato prorogato il credito di imposta sugli affitti anche alle attività di imprese con fatturato superiore a 15 milioni e situate nei centri commerciali. Alcuni temi sono ovviamente rimasti irrisolti e aperti e qualche ordine del giorno è stato da noi presentato anche in questa sede. In particolare,

la possibilità di cedere il credito di imposta. Questo è fondamentale. *(Applausi)*. Le questioni aperte, dunque, sono ancora molte, ma la Lega continuerà a proporre soluzioni concrete e sarà sempre a fianco delle aziende e delle persone che lavorano. sostegni *bis* è arrivato in Senato nella prossimità della scadenza e quindi è stato esaminato in modo molto rapido: non abbiamo avuto la possibilità di esaminarlo in modo approfondito e soprattutto di proporre e di approvare delle modifiche.

che interessano gli uffici legislativi di tutti i Ministeri e del Parlamento. Su questo dovremmo interrogarci, nel senso che dovremmo trovare la formula adatta, corretta e idonea, per fare in modo che i provvedimenti vengano esaminati in modo concreto da entrambi i rami

i senatori e i deputati hanno il diritto di proporre delle modifiche a tali provvedimenti, ma purtroppo la poderosità e l'ampiezza di questi strumenti è così elevata,

che ci costringe a questo bicameralismo a senso unico alternato, ma non è una critica da fare al Governo, perché purtroppo dobbiamo renderci conto del fatto che la nostra struttura non è abituata ad esaminare

quelli che volevano costruirsi una famiglia. Adesso invece si fa un passo indietro, che per fortuna durante l'*iter* parlamentare alla Camera dei deputati è stato comunque rivisto. È stata infatti aggiunta una clausola in più e una causale in più, certo discussa a livello di contrattazione nazionale collettiva,

e dico che il *cashback* è una misura che è servita molto. È servita perché 9 milioni di cittadini italiani, grazie al *cashback*, hanno deciso di installare l'applicazione IO. In questo periodo le applicazioni sono molto importanti, perché permettono, soprattutto l'*app* IO, di creare un'interfaccia tra cittadino e Stato, tra cittadino e pubblica amministrazione, tra cittadino e servizi di cui devono godere i nostri cittadini. Senza queste applicazioni, questi servizi non vengono utilizzati; quindi è utile migliorare il dialogo, migliorare la *compliance* tra cittadini e pubblica amministrazione e fare in modo che sia più semplice interagire. Visto che chiediamo spesso

la famosa evasione fiscale, di cui ci lamentiamo spesso, dicendo che va combattuta. L'*app* IO, e soprattutto il *cashback*, consentono di ridurre l'evasione fiscale, perché le operazioni vengono premiate se sono tracciate e se vengono utilizzati strumenti tracciabili, come ad esempio la moneta elettronica. Quindi il *cashback* è servito,

Siamo riusciti - perché parlo come Parlamento - a ridurre l'IVA sulle bestie vive e sugli animali vivi utilizzati come richiami per la caccia. Già si tratta di una barbarie; ora noi andiamo pure a incentivare questa barbarie.

Vi è un altro provvedimento, fortemente voluto da un Gruppo di questo Senato e della Camera, che riguarda le sigarette elettroniche. Anche in questo caso era stato dichiarato inammissibile al Senato, ma è stato proposto alla Camera ed è stato approvato. Ora, la tassazione sulle sigarette elettroniche è una questione molto delicata, perché le sigarette elettroniche contengono anche la nicotina; andare a toccare la tassa sui prodotti che contengono nicotina può influenzare i consumatori, ma non attraverso il *marketing*, bensì attraverso il fatto che comunque assumono nicotina. Quindi non è detto che abbassando la tassa si abbia un maggiore consumo di sigarette elettroniche; potrebbe crescere anche il consumo di sigarette vere e proprie, perché contengono nicotina anche le sigarette normali. Questa è una misura molto delicata, che avrebbe dovuto essere adottata in un provvedimento a sé; invece è stata introdotta in questo decreto-legge sostegni, sempre con la scusa della pandemia. Ma non solo: questo provvedimento di riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche arriva dopo altri favori fatti ai produttori e ai distributori di sigarette elettroniche nel 2018, quando la tassa era stata abbassata del 95

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi)*.

i giornali della Sardegna, e in modo particolare del Sulcis,

Una persona sta male, un elicottero la soccorre e la porta sulla terraferma; atterra in un campo sportivo, lo stadio di Carbonia,

e nessuno apre la porta dello stadio. I vigili del Comune di Carbonia arrivano abbondantemente in ritardo - si parla non di cinque o dieci minuti, ma molto di più - e la persona

e non apre le porte dello stadio, del campo sportivo, dove una persona sta male e sta aspettando di essere soccorsa dall'ambulanza.

e di aver provocato la morte di una persona. Signor Presidente, ricorre oggi il ventesimo anniversario di accadimenti sconvolgenti che rappresentano una pagina nerissima per la nostra Repubblica: pagina ricordata come «la notte della macelleria messicana» - come la definì il vice questore Michelangelo Fournier - o come la più grande sospensione della democrazia e dei diritti civili dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il 21 luglio del 2001, in occasione del G8 a Genova, dopo una giornata drammatica, le Forze dell'ordine fecero irruzione alla scuola Diaz-Pertini a Genova per quella che doveva essere una perquisizione e che invece degenerò in una sorta di spedizione punitiva per i manifestanti pacifici e per i giornalisti che erano lì

come del resto accadde a tutti quelli che erano appunto all'interno della scuola. Gli intollerabili atti di tortura e di umiliazione continuarono alla caserma Molti esponenti delle Forze dell'ordine sono riusciti a sfuggire alla giustizia, non essendo riconoscibili, e a tal proposito l'Unione europea aveva raccomandato a tutti i Paesi dell'Unione di dotare le Forze dell'ordine di elementi identificativi. A questa raccomandazione hanno poi adempiuto adempiuto ben 20 Paesi sugli allora 28, ma purtroppo l'Italia non ha mai accettato questo invito. Anzi, alcuni esponenti, peraltro apicali, sono stati riconosciuti colpevoli, ma le condanne non sono state scontate anche per via dell'indulto. Dirò di più: nessuno dei condannati ha avuto problemi di carriera ed alcuni hanno anche assunto delle cariche importantissime, come se avessero ricevuto un premio.

quello energivoro, che ha effetti nefasti sull'ambiente; se fosse giusto adottare una globalizzazione selvaggia che causava enormi squilibri territoriali e ambientali, nonché ingiustizia sociale, o perseguire quello che proponevano i Paesi del G8

non si verifichino più e auspichiamo che l'Italia si doti di una legge contro la tortura, che dia la possibilità di identificare gli esponenti delle Forze dell'ordine, proprio a garanzia dei tanti dei tanti - sono la stragrande maggioranza - uomini e donne delle nostre forze di polizia che svolgono con competenza, amore e professionalità il proprio lavoro. Lo dobbiamo a loro Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la Commissione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione ha recentemente approvato le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 ed è notizia di qualche giorno fa l'approvazione dell'intesa in Conferenza unificata Il testo delle linee pedagogiche è stato sottoposto a un'ampia azione di informazione e consultazione pubblica prima di arrivare alla stesura finale. Secondo il Ministero rappresenta una cornice di riferimento pedagogico e il quadro istituzionale organizzativo in cui si colloca il sistema educativo integrato. Qualche giorno fa l'Associazione dei pedagogisti educatori italiani (APEI) ha inviato una missiva al Ministro dell'istruzione evidenziando l'importanza di un approccio pedagogico nel contesto dell'educazione per tutto il segmento di età da zero a sei anni, sostenendo proprio la necessità di inserire nei ruoli professionali, a fianco di bambine e bambini, i professionisti dell'educazione. Ritengo sia indispensabile che il Ministero faccia proprie tali proposte nello sviluppo del sistema integrato, assicurando un pieno riconoscimento del contributo delle professioni pedagogiche attraverso la scelta del loro utilizzo per tutto il segmento 0-6. Ciò in quanto i laureati in ambito pedagogico sono i professionisti più in grado di saper rispondere con consapevolezza e competenza alle esigenze educative dei bambini e delle bambine. Per tali ragioni è opportuno inserire la figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia non solo nei nidi, ma anche nella scuola dell'infanzia, in quanto l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che lavora con tutte le età della vita da zero a sei anni, è laureato in scienze dell'educazione e della formazione. Al contempo è necessario affidare il coordinamento pedagogico dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia alla figura del pedagogista, il quale rappresenta il più grande esperto di educazione infantile, essendo proprio conoscitore dei processi di sviluppo dei bambini. La figura del pedagogista appare anche quella più consona all'affidamento della funzione di promozione e valorizzazione delle competenze genitoriali. Se, dunque, era già necessario l'inserimento a regime di tale figura, lo è ancora di più in questo periodo di emergenza epidemiologica, in quanto c'è il rischio di conseguenze nefaste per lo sviluppo della personalità umana. Se negli ultimi anni si è giunti a un livello di riflessione e consapevolezza sul tema dell'educazione prescolare

e pedagogisti, figure i cui percorsi di studio si pongono l'una in linea di continuità con l'altra, anche in affinità ai percorsi formativi degli insegnanti della scuola dell'infanzia, raggiungere l'obiettivo prefigurato risulterebbe ben più arduo e difficoltoso, anche nell'ottica della migliore spesa delle risorse stanziate, che ammontano a 309 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2021-2025.

alle RSA. L'8 maggio di quest'anno è stata approvata un'ordinanza di accesso familiari e visitatori da parte del Ministero della salute. In detta ordinanza, purtroppo, è rimasta tutta una serie di incertezze interpretative, legate alle disponibilità di personale e alle condizioni favorevoli, che, di fatto, hanno scaricato gran parte delle decisioni sulle spalle del direttore sanitario delle strutture. Questo ha comportato, nella maggior parte delle strutture, una scarsa disponibilità all'apertura agli ospiti, visitatori e familiari. Dato che detta ordinanza è in scadenza alla fine di luglio del corrente mese, sono a richiamare, cogliendo a pretesto proprio l'interrogazione cui facevo riferimento prima, il Ministero della salute a emanare, nella nuova ordinanza, definizioni più puntuali, che non scarichino sulla valutazione da parte del direttore sanitario delle condizioni di contesto. Questo porterà come è successo negli ultimi mesi - a una ampiamente difforme applicazione dell'ordinanza nelle varie strutture e, in molti casi, a ragionare più a tutela più a tutela della struttura che non sulle finalità dell'ordinanza, e cioè stabilire condizioni e regole per l'accesso di familiari e visitatori alle strutture. Questo anche in un'ottica di benessere complessivo degli ospiti delle stesse.